avevate promesso alle famiglie - che hanno bevuto le vostre frottole in campagna elettorale - meno tasse e più sviluppo, meno burocrazia e più concorrenza, trasparenza negli atti di Governo, legalità per mettere alle spalle il vecchiume della Prima Repubblica; promesso che, a differenza del precedente Governo, non avreste mai messo le mani nelle tasche degli italiani. Tuttavia, è dal maggio 2008, da quando avete ricevuto la fiducia da una maggioranza blindata, mai vista prima nei due rami del Parlamento e che scricchiola ogni giorno di più - e per questo chiederete il 34° voto di fiducia che avete cominciato ad introdurre tutta una serie di tributi, tasse, balzelli, pedaggiamenti, rincari, ritocchi, stangate per i comuni cittadini e tagli agli stipendi, ai salari e alle pensioni dei vecchi, suffragati da politiche di condoni, perdoni, scudi per le *élites* mai visti prima nella storia di Repubblica. Invece degli sgravi fiscali e degli aiuti alle famiglie, dei rimborsi agli azionisti di Alitalia e al popolo truffato dalle banche, della trasparenza e della concorrenza, avete assecondato le varie cricche di potere, gli appalti senza gare, gli scandali del G8 e della Maddalena, dell'eolico e di una Protezione civile che ha agito al di fuori della legalità per far conseguire traffici ed affari ai soliti che pregustavano sotto le lenzuola i fiorenti appalti della ricostruzione dell'Aquila. Tra tariffe aeroportuali per assecondare i capitalisti dei pedaggi (come il dottor Palenzona di Unicredit-Aiscat), pedaggiamenti ANAS, rincari delle tariffe elettriche e del gas, ritocchi dei servizi idrici, aumenti dei biglietti dei treni - dove avete voluto sistemare in una comoda poltrona di prima classe una cariatide, che risponde al nome di Lamberto Cardia, come diretta ricompensa per i servigi svolti a vostro favore tariffe sui rifiuti, addizionali locali, mancati trasferimenti agli enti locali e la riesumazione dell'ICI, voi, signori del Governo, avete messo tutte e due le mani nelle tasche delle famiglie, con un costo annuo pari a 886 euro. Alle imprese di assicurazione avete applicato il minimo sindacale, ma non avete neppure sfiorato nella manovra i signori del credito e quei capitalisti delle bollette e dei pedaggi che vessano ogni giorno i cittadini. La politica economica degli ultimi due anni è fallimentare: oltre ad aver prodotto un aumento del debito pubblico - passato dai 1.663 miliardi di euro dell'aprile 2008 ai 1.827 miliardi di oggi (il riferimento è al maggio scorso), con un aumento di 164 miliardi di euro - con la politica di condoni e perdoni fiscali, previdenziali, ambientali, esattoriali ed il varo della più grande operazione di riciclaggio di Stato, come deve essere definito lo scudo fiscale "criminale" con la sua forma anonima di rientro dei capitali, avete generato una disaffezione dagli obblighi fiscali, posto che sarebbe stata legittima difesa il mancato pagamento di tasse, con un'evasione fiscale che ha raggiunto 120 miliardi di euro. Il Governo, pur annunciando propositi liberisti, non ha promosso il mercato e la concorrenza, ma, al contrario, ha smantellato le liberalizzazioni dell'ex ministro Bersani; ha svuotato di contenuto la *class action* come utile strumento di deterrenza in mano ai cittadini verso i comportamenti fraudolenti dei manutengoli del potere economico; sanato con leggi *ad hoc* le condotte scorrette e vessatorie delle banche (mi riferisco alla commissione di massimo scoperto, agli *swap* e ai derivati appioppati agli enti locali per oltre 30 miliardi di euro ed alle piccole e medie imprese portate al fallimento). Monopoli, oligopoli e cartelli operanti in settori al riparo della concorrenza possono brindare per questa manovra e quasi tutti i soggetti che hanno avuto la possibilità di determinare prezzi e tariffe hanno avuto mano libera per aumentarli,

La ricetta per far ripartire i consumi incitando le famiglie ad indebitarsi con la cessione del quinto dello stipendio dei lavoratori privati, atipici e pensionati, le offerte di pagamenti rateizzati, i cosiddetti prestiti vitalizi per far ipotecare le case dei vecchi, invece di far leva sulla creazione di ricchezza derivante dalle liberalizzazioni e dal mercato, con una distribuzione di maggiori redditi mediante l'abbattimento dei prezzi, l'eliminazione delle strozzature del mercato (come le rendite di posizione) e la liberalizzazione delle professioni e di alcuni mercati protetti (aeroporti, autostrade), hanno mostrato tutta la loro debolezza ed inefficacia. Sulla gravissima crisi della Grecia Goldman Sachs - che all'epoca annoverava come vice presidente per l'Europa che aveva appaltato, come direttore generale del Tesoro, importanti privatizzazioni alla banca d'affari sul famoso panfilo Britannia - è accusata di aver svolto un ruolo importante. Secondo singolari teorie rappresentate dai *mass media*, le banche italiane, più virtuose delle altre, avrebbero sofferto meno gli effetti della crisi sistemica. Ma giova ricordare che le virtuose banche italiane, ben protette dalla Banca d'Italia, che vede tra

cento in più rispetto all'Europa. E mentre il procuratore di Milano Robledo ha sottoposto a processo alcune banche per la vendita di derivati al Comune di Milano e ha messo in guardia sul rischio della bomba derivati sugli enti locali (pari ad oltre 30 miliardi), la Banca d'Italia, a lungo distratta, comincia a pubblicare i dati sui *credit* *default* *swap* (CDS) detenuti dagli istituti di credito italiani, che al 31 dicembre avevano una consistenza di 762,3 miliardi di euro.

Questa è una manovra del tutto insufficiente, rispetto agli 80‑100 miliardi di Francia e Germania, che fa gravare i costi della crisi soprattutto sulla povera gente. Invece si poteva agire

si potevano introdurre un'aliquota del 3 per cento sulla commissione di massimo scoperto e un'imposizione fiscale dell'1,5 per cento sulle transazioni in CDS.

caste popolate da pseudo-autorità sedicenti indipendenti, che non rispondono ad alcuno del loro operato, con la licenza di intrallazzi, clienti, sprechi, privilegi. Non mi dilungo sulla scandalosa ISVAP, su una CONSOB adusa ad assunzioni clientelari di figli e parenti di papaveri, senza concorsi pubblici e per chiamata diretta, con successive dorate carriere pilotate da concorsi interni. Non mi dilungo sulla AGCOM, che potrebbe essere accorpata sull'esempio della FSA inglese, per offrire maggiore efficienza ed un grado accettabile di concorrenza e di sana trasparenza. Vado ad una proposta, quella della Banca d'Italia. La tavola 22.1 della relazione annuale, diffusa il 31 maggio, illustra la composizione del personale: 653 dirigenti, 1.450 funzionari, 1.273 coadiutori, 4.147 altro personale. A pagina 306 della relazione, nella tabella del conto economico, si leggono dati eclatanti sugli stipendi, di questa cricca che non ha vigilato sui mercati. Questi signori costano 1,3 miliardi di euro. Tenere in piedi una Banca d'Italia che non ha mai tutelato i diritti dei risparmiatori e consumatori, ma ha sempre difeso gli interessi predatori delle banche, con tassi più elevati e condizioni più onerose e con i costi di gestione più alti al mondo dei conti correnti

si gode di trasferte di 300 euro per andare a lavorare a Roma. Come se fosse una grande impresa, Bankitalia ha attivato un servizio di attività immobiliari di circa 300 persone, delle quali 50 effettuano quattro missioni al mese,

Oltre ai servizi tecnici, per le gestione del patrimonio immobiliare di Roma, esiste una società al cui vertice è stato collocato il dottor Scimia, ex funzionario generale. C'è poi il CASC (Centro per l'assistenza sociale e culturale), occupa un convento al Mandrione, all'interno di un grande parco su quattro piani di circa 1.000 metri quadri, il cui restauro è costato 6 milioni di euro, ed è gestito da un consiglio e da un presidente eletto dai sindacati, che in occasione delle votazioni si accapigliano per gestire un affare miliardario: la Banca fornisce 30 dipendenti. Addirittura, si tengono all'estero tornei di *bridge* e di scopetta, sulla pelle della povera gente e dei pensionati. La GIAFI Costruzioni, che ha l'appalto della manutenzione a Roma della Banca d'Italia, è nell'elenco delle società che hanno partecipato ai lavori per il G8 alla Maddalena. Nell'ambito della politica di bilancio restrittiva, è scandaloso che il Governatore della Banca d'Italia continui a chiedere al Paese e agli italiani sacrifici, mentre il personale dell'Istituto è pieno di privilegi. Ripeto: 653 dirigenti e 1.450 funzionari

generata dall'avidità dei banchieri e dalle collusioni delle attività di autorità di vigilanza distratte, si doveva evitare che a pagare fossero i soliti lavoratori e pensionati, esentando sedicenti autorità indipendenti che come loro principale *mission* hanno il perseguimento dei privilegi, non gli interessi generali del Paese. la politica ha concesso generose deleghe in bianco a una classe di oligarchi che, oltre a non rispondere ad alcuno del proprio operato, è adusa ad agire nell'ombra e nell'opacità per difendere privilegi di casta, tramando sottobanco contro gli interessi generali, con l'esclusiva finalità di tutelare se stessa e un sistema bancario paramafioso, cui è legata a doppio filo, e che ha provocato disastri e continuerà a produrli, se non vengono prese immediate contromisure. Perché non le si presenta mai il conto, signor Presidente, colleghi? Perché non si recidono sperperi sprechi, clientele, favoritismi inaccettabili, regalie, forse perfino atti di corruzione all'interno di un sepolcro imbiancato? Gli ispettori della Banca d'Italia guadagnano

Addirittura, quando escono dalle ispezioni, si ritrovano anche assunzioni nelle casse e nelle banche ispezionate, perfino dei loro camerieri. di un sepolcro imbiancato rispetto al quale fino a ieri era vietato ai rappresentanti del popolo perfino di porre domande ed interrogativi con gli strumenti del sindacato ispettivo. La casta delle caste, denominata Bankitalia, che cogestisce assieme ai sindacati 1,3 miliardi di euro l'anno tra stipendi, prebende e spese di amministrazione tanto riservati quanto bui ed insindacabili, con semplici ispettori che - lo ripeto - arrivano a guadagnare 580.000 euro l'anno, il quadruplo di un parlamentare, ricevendo dalle casse e banche ispezionate favori ed assunzioni clientelari, deve cominciare a rispondere del suo scandaloso operato. Ma di questo non c'è traccia nella manovra. Voi, signori del Governo e signori della maggioranza, siete forti con la povera gente, con i deboli - avete fatto picchiare pure i terremotati dell'Aquila - ma siete deboli con il grande potere. Mi auguro che prima o poi si debba rendere conto di quello che accade. Solo così si rende un servizio ai cittadini, toccando la casta delle caste, scoperchiando le malefatte, e si renderà un servizio agli interessi generali del Paese ed ai lavoratori che sono licenziati e pagano i costi della crisi per precise responsabilità, che hanno nome e cognome: banchieri d'affari, banche, autorità vigilanti.

dovrò, mio malgrado, rinunciare a sviluppare alcune considerazioni tra la politica ed il folklore. Vorrei però lasciare in non ai colleghi della maggioranza, che sono desolatamente assenti, ma almeno al Resoconto stenografico, alcune valutazioni che ritengo debbano pur sempre essere svolte. Desidero affermare, senza alcun tentennamento, che la manovra che stiamo discutendo, a nostro giudizio, non corrisponde assolutamente alle caratteristiche che sono state aulicamente illustrate dal ministro Tremonti, il quale ha detto - sempre più convinto del fatto che il popolo italiano sia totalmente privo di qualunque capacità di discernimento

L'affidabilità e l'attendibilità di queste affermazioni corrispondono direttamente all'attendibilità che ha il PdL quando si propone come partito dell'amore,

in Parlamento, ancorché in un'Aula semideserta, il Partito Democratico desidera chiarire agli interlocutori virtuali, - cioè coloro che possono leggere gli atti parlamentari o seguire le trasmissioni - che non abbiamo bevuto nessuna di queste frottole, di questo campionario di insulti all'intelligenza del popolo italiano che ci viene regolarmente propinato. propinato. Nei pochi minuti che mi rimangono svolgerò alcune considerazioni relativamente al comparto difesa e sicurezza per fare delle constatazioni alle quali seguiranno delle affermazioni. Due anni fa questa maggioranza ha vinto le elezioni politiche, prevalentemente facendo leva sul valore anche etico e non solo politico della sicurezza. Ha creato condizioni di paura, ha alimentato in certi casi anche il terrore, ha creato un bisogno di tranquillità e di sicurezza, usando una retorica di antica memoria nei confronti degli uomini della legge. Oggi, quasi a conclusione della seduta antimeridiana, c'è stato un applauso scrosciante che ha salutato la comunicazione fatta dal Presidente del Senato a proposito di una serie di arresti

non soltanto con le donne e gli uomini in uniforme, ma anche con quelli che lavorano nelle strade. Ebbene, anche questa è tutta una finzione, una drammatica, terribile, scandalosa presa in giro, perché nei confronti di questi 550.000 italiani si sta consumando un atto di ingiustizia che non ha eguali nella storia democratica.

tanto che il Capo di Stato maggiore della Difesa ha affermato che il grado di addestramento dei nostri militari non è tale da offrire le necessarie e giuste garanzie per un impegno nei teatri internazionali.

la condizione operativa sia dei soldati che delle forze dell'ordine. Ci sarà però la mini-naja,

si sarebbero invece potuti finanziare ben 6.000 militari veri, che anziché essere stabilizzati nel loro lavoro, dovranno lasciarlo. Dopo Dopo essere stati impegnati per sei anni al servizio del nostro Paese, trascorrendo magari anche due anni in Afghanistan o in altri teatri internazionali di guerra, vengono mandati via, perché sono più importanti

un Paese serio e civile, un Governo che meriti di guidare una Nazione come la nostra non si sognerebbe mai di cadere in questo tipo di atteggiamento. dunque che ci sia un sussulto di dignità, che i nostri emendamenti vengano esaminati, che non si ricorra al voto di fiducia e che si abbia, almeno una volta in due anni ‑ in fondo non è poi così tanto la bontà, la correttezza e la cortesia di trattare gli italiani come un popolo civile e non come qualcosa di diverso.

Quindi, per fortuna, grazie a quelle capacità previsionale, oggi ci troviamo a vivere questo momento, delicato per tutti ad ogni livello,

signor Presidente, signor rappresentante del Governo, gentili amici e colleghi

il 19 marzo 2009 il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, esprimeva alla Commissione finanze della Camera il suo parere sulla crisi in corso (mi dispiace che non ci sia il collega Lannutti, avrei tante cose da rispondergli, ma si vede che è dovuto andare via). In quell'occasione, il Governatore riconosceva un gran numero di positività nell'azione del Governo: tra queste, il Fondo per garantire il sostegno delle banche alle piccole e medie imprese; i meccanismi temporanei di sostegno al reddito per i dipendenti di imprese non protette dalla cassa integrazione guadagni; le misure di sostegno alle imprese attraverso interventi in corso di definizione con la Cassa depositi e prestiti e la SACE; il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio dei costi standard (novità importantissima e basilare per ogni settore). Il Governatore terminava la prima parte del suo discorso dicendo: «In paesi come l'Italia, dove è alto il debito pubblico, interventi di breve periodo ampi e incisivi vanno compensati da misure strutturali che diano subito la certezza del riequilibrio del bilancio nel medio periodo. Allungare lo sguardo è essenziale: la sostenibilità dei conti pubblici nel lungo periodo è fondamentale anche per assicurare l'efficacia delle politiche di breve». Il rapporto sistemico tra le politiche economiche di breve periodo, comprese quelle monetarie, e l'equilibrio dei conti economici del Paese è, se possibile, oggi ancora Ci viene portato, come motivazione contraria alla manovra, il fatto che essa avrà un effetto recessivo sulla timida ripresa dell'economia reale oggi in corso (già è in corso una timida ripresa: è già qualcosa). È vero, lo sanno tutti, la manovra avrà un impatto negativo sul PIL dello 0,5

Il solo modo per neutralizzare tale effetto era di rendere più competitive le nostre esportazioni con un'azione di riequilibrio del rapporto di cambio euro-dollaro, cosa che è avvenuta (ricordiamoci quanto era quotato il dollaro rispetto all'euro qualche tempo fa).

cinese rende oggi la Cina un mercato dove esportare, non solo un'area dove produrre a basso costo; questo forse gli italiani dovrebbero Ciò consentirà anche di recuperare l'effetto depressivo della manovra in quei Paesi le cui imprese sapranno approfittare della contingenza monetaria favorevole. La vera sfida, dunque, è mettere le nostre imprese in grado di competere sui mercati internazionali. In questo disegno dobbiamo riconoscere al *premier* Berlusconi, che nei giorni scorsi ha fatto il giro di mezzo mondo per procurare miliardi di commesse per il lavoro italiano all'estero, di essere l'elemento di traino per il Paese. Invito poi la sinistra a non proporre politiche di espansione della domanda interna: con il terzo deficit pubblico più alto del mondo - è inutile che lo ricordiamo - rischieremmo di vedere fallire il nostro Stato, che già adesso fatica a piazzare i titoli per finanziare il proprio debito. Nel merito, la manovra vorrebbe colpire gli sprechi ed essere solo giusta, tagliando gli sprechi e spingendo l'economia, per consentire la ripresa del tessuto economico e sociale nel nostro Paese, cioè far tornare il livello di vita degli italiani in un contesto che non sia al di sopra delle loro possibilità.

Province. Malgrado quello che ha scritto «l'Unità» a proposito di sprechi, la manovra non è spietata con gli invalidi, recupera effetti particolarmente negativi per il personale della scuola

Un discorso a parte merita il nuovo progetto pensionistico introdotto dall'emendamento governativo che, giustamente, conserva il diritto maturato alla pensione per chi ha 40 anni di contributi. La pensione è un diritto, non un regalo dello Stato! Anticipare l'elevazione dell'età pensionabile, collegandola all'allungamento delle aspettative di vita è una piccola rivoluzione che tiene conto del miglioramento della qualità della vita e che consente di avvertire come un'opportunità il prolungato mantenimento sul posto di lavoro.

a quelle donne - le casalinghe - di cui nessuno parla: donne che devono lavorare per affermarsi, che scelgono di restare in casa a curare i figli o gli anziani non autosufficienti o a dedicarsi alla propria famiglia, e che costituiscono gran parte di quel tessuto sociale e relazionale che forma la nostra comunità. Occorre, onorevoli colleghe e colleghi, iniziare ad affrontare questo problema. Non è accettabile che lavoratrici, come le casalinghe, non abbiano una pensione, che nessuno pensi a loro, e che a 65 anni debbono ancora chiedere i soldi al marito. Questo è vergognoso. Mi chiedo, infine,

A questo proposito rilevo che le possibilità di scegliere in maniera più ragionata sono state poche. Auspico dunque che almeno gli enti di ricerca e formazione indispensabili, come per esempio l'ISPESL,

Si colpiscono le consulenze, è vero, e i costi di rappresentanza, ma nessun dipendente perde la propria qualifica o viene licenziato, nemmeno negli enti che spariscono o sono accorpati.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, è davvero un peccato, oltre che un grave limite per la democrazia, il fatto che, ancora una volta, il Governo si sia voluto sottrarre alla possibilità di un confronto concedere la possibilità, a tutto il Parlamento, di fornire utili contributi per migliorare e qualificare meglio la manovra che arriva in Aula. Purtroppo il Governo ha deciso, e reiteratamente lo ha fatto in questi due anni, di ridurre il Parlamento a luogo di mere ratifiche, esautorandolo per l'ennesima volta dei suoi poteri. Ma questo Governo è stato, in questa fase e in questa vicenda, sordo non soltanto al Parlamento, ma anche a tutto il sistema delle autonomie territoriali. Pensiamo, per esempio, allo scontro intervenuto con le Regioni, che è anche sintomatico di chi ha deciso d'imporre prove di forza per coprire, evidentemente, la propria debolezza e la propria fragilità. La collega che mi ha preceduto ha giustamente sottolineato che questa è una manovra necessaria e che il Paese deve porre in sicurezza i conti pubblici. È una manovra fatta anche in altri Paesi, anche in Paesi dall'economia più florida della nostra. In questi Paesi, però, i Governi si sono posti un duplice un duplice obiettivo: quello d'imporre i sacrifici, sicuramente, e di fare tagli, ma anche l'obiettivo di fare investimenti di aiutare le giovani generazioni. Questa manovra, invece, (una manovra imponente, pari a quasi 25 miliardi di euro) non è stata accompagnata da alcuna significativa misura per il sostegno della domanda e dell'offerta; non ha definito nessun obiettivo strategico sul terreno della ripresa economica e nessuna delle priorità del Paese viene in essa affrontata: la crescita della disoccupazione, disoccupazione, le difficoltà del tessuto imprenditoriale e la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro e pensione. Non sono previste misure per il sostegno del settore del turismo,

con questa manovra il Mezzogiorno, per il quale si profila un'altra pesante sottrazione di risorse. Con essa sfuma qualsiasi possibilità di intraprendere e portare a termine un qualsiasi progetto di moderno e serio sviluppo di quelle aree, momento che, per ogni esigenza di copertura, la parola d'ordine del Governo è di utilizzare i fondi FAS: come un bancomat infinito, presidente Azzollini, destinato agli interventi più diversi, ma del tutto estranei al riequilibrio socio-economico del Mezzogiorno.

meridionalista. Anzi, i provvedimenti fin qui varati, non ultima la finanziaria 2010, hanno di fatto azzerato ogni intervento a favore del Mezzogiorno e del suo sviluppo e permesso il continuo ricorso al FAS nazionale per la copertura di provvedimenti di carattere generale. generale. Questa sistematica distrazione di fondi, valutabile nella somma di circa 35 miliardi di euro, compromette non solo il rispetto dell'originario vincolo di ripartizione delle risorse del Fondo, ma di fatto azzera le politiche di sviluppo che le Regioni del Sud realizzano

Il Governo non ha mai posto fine a questa dilapidazione. Adesso il ministro Tremonti accusa le Regioni meridionali di cialtroneria per la lentezza con cui spendono i fondi comunitari loro assegnati. Ben vengano le osservazioni a chi ha fatto degli errori, ben vengano le critiche costruttive, ma innanzitutto si faccia un'operazione di chiarezza e si spieghi per cosa sono stati utilizzati i fondi FAS:

annunciato più di un anno fa dal non rimpianto ministro Scajola come decisivo e innovativo. Che fine ha fatto quel piano? Che fine ha fatto la Banca per il Sud? Che fine hanno fatto le risorse del FAS? Perché per registrare una delibera del CIPE ci vuole più di un anno? È da un anno, infatti, che si aspetta la pubblicazione della delibera 51 del 26 giugno 2009 che ripartisce le risorse del Fondo.

per un'autostrada che non è stata mai finita. Sull'abolizione delle zone franche, in realtà il Governo è stato coerente. Sono due anni che cerca di abolire le zone franche e lo ha fatto, sostituendole con delle zone a burocrazia zero

vorrei esordire con una manifestazione di stupore e di disappunto perché tutti gli emendamenti da me presentati, finalizzati all'incremento delle entrate, e nonostante i buoni uffici del presidente Azzollini, hanno avuto parere contrario da parte del Governo, a partire da quell'emendamento, essenziale per una democrazia vera e non formale, che prevede l'abolizione di tutti i privilegi per tutte le cariche pubbliche,

non può mantenere benefici e privilegi alla cessazione della carica; non è accettabile che i Presidenti di Camera e Senato alla fine del loro mandato studino quale ufficio, quali appartamenti, quali benefici e servigi debbano mantenere. Quindi, che l'esempio venga dall'alto e non dal basso Io ripresenterò questo emendamento in tutti i provvedimenti che il Governo sottoporrà al Parlamento fino alla fine della legislatura. Va dato atto al Governo Berlusconi e al ministro Tremonti di aver mostrato coraggio e determinazione nel proporre questa brusca manovra correttiva delle inquietanti tendenze dei conti pubblici, benché sarebbe stato meno doloroso per il Paese se l'azione di contenimento fosse stata portata avanti progressivamente fin dai primi anni di questo decennio. la bontà di una manovra di riduzione del disavanzo su base pluriennale si misura essenzialmente dalla capacità di raggiungere i traguardi prestabiliti e di minimizzare nel contempo il danno collaterale sul versante della crescita economica. Se le misure di riduzione della spesa e di incremento delle entrate deprimono la formazione del reddito, il risultato atteso potrebbe essere mancato perché non si raggiunge l'obiettivo di abbassare il rapporto tra deficit e PIL nella quantità desiderata; bisogna in altri termini fare attenzione a quali poste vanno tagliate e quali vanno preservate per non essere costretti in seguito a una nuova e dolorosa correzione per raggiungere il prestabilito rapporto *deficit*-PIL. In particolare, se i tagli operati sulla spesa deprimono gravemente la crescita economica, dato che questa influisce a sua volta sul gettito fiscale, l'effetto finale potrebbe essere di non riuscire a realizzare grandi progressi nella direzione auspicata. Parimenti, se questa manovra non conduce per diversi anni a un consistente avanzo primario nel bilancio, non è tecnicamente possibile a parità di altre condizioni, incluso l'atteggiamento della politica monetaria - riportare il rapporto debito-PIL sotto il limite di sicurezza del 100 esaminati i 56 articoli del provvedimento, si avverte chiaramente che il rigore non sembra accompagnarsi alla creazione di nuove consistenti opportunità di espansione economica, né per le imprese né per le famiglie. Di fronte a tagli della spesa pari allo 0,8 per cento del PIL per ciascun anno del prossimo di biennio, le possibilità di migliorare la crescita stabilmente dipendono essenzialmente da tre condizioni: la scelta di ridurre le poste a minore impatto sullo sviluppo, lasciando più spazio alle altre; il riorentamento delle risorse verso gli investimenti fissi; l'impulso al miglioramento della redditività e competitività delle imprese, lasciando da parte i guadagni effimeri di mercato dovuti al forte deprezzamento dell'euro. Bisogna puntare, in breve, su una maggiore qualità della spesa pubblica e sull'alleggerimento della fiscalità sulle imprese. Sotto questi profili la manovra in esame lascia a desiderare, perché taglia gli investimenti più che la spesa corrente, né offre alle imprese impulsi ad espandere la produzione e a creare nuova occupazione a compensazione di quella che verrebbe distrutta nel settore pubblico. Ne è riprova il fatto che attualmente la ripresa dell'attività produttiva è trainata essenzialmente dagli ordinativi esteri, in parte gonfiati dal recente deprezzamento dell'euro. Ma un giudizio definitivo sulla manovra non si può dare, perché essa presenta oggi grandi aree di incertezza nei suoi effetti quantitativi di riduzione di spese e incrementi di entrate, come riconosciuto nella stessa Relazione tecnica in diversi punti. Molto del risultato dipenderà dal modo in cui sarà gestita. Pertanto, l'approvazione del provvedimento in sede parlamentare di fatto è una delega a correggere i conti in misura non pienamente determinata *a priori*. La soppressione di alcuni enti dà risparmi modesti, per via dell'assorbimento del personale relativo, mentre provoca discontinuità nell'operare della pubblica amministrazione. La spesa in conto capitale, tra cui quella per investimenti, verrebbe ridotta del 5,5 per cento nel prossimo biennio, una diminuzione che, per via dei suoi effetti demoltiplicativi sulla domanda interna, incide sul potenziale di sviluppo futuro dell'economia e forse sulla competitività sistemica, se tocca spese infrastrutturali. L'occupazione è giustamente obbligata a ridursi nel settore pubblico, ma quali nuove possibilità di impiego si creerebbero nel privato per le forze di lavoro disoccupate, se per le imprese la manovra non contiene misure per innalzare la redditività degli investimenti, ad esempio, attraverso o una minore tassazione o un'offerta da parte del soggetto pubblico di maggiori economie esterne di sistema? I benefici fiscali per i contratti di produttività servono poco allo scopo, soprattutto quando in prospettiva vi è una stasi della domanda interna, perché mirano a migliorare la produttività, non ad ampliare la platea degli occupati. Le reti di imprese dovrebbero godere di alcuni benefici, ma non sono specificati quali e quanti; in ogni caso sarebbero di modesto impatto. La deburocratizzazione di alcune zone del Meridione è molto utile, ma soggetta a diverse condizioni che ne possono limitare la portata. Il Sud è colpito dalla manovra come le altre aree del Paese, nonostante la fiscalità di vantaggio possibile per l'area. Questa è una possibilità, non una certezza, considerato che le Regioni, che già vedono decurtati i trasferimenti dallo Stato, devono reperire le necessarie risorse, prelevandole da altri capitoli di spesa. Per altro verso, le risorse del FAS destinate al Mezzogiorno, dopo il loro parziale dirottamento verso altri scopi, non sono state ripristinate ai livelli iniziali. Sarebbe invece auspicabile e necessario per questa zona, che ha sofferto maggiormente nella recessione, poter contare su più efficaci misure di rilancio della crescita. Sul versante delle entrate, è positivo che non vi siano sostanziali aggravi e che si intensifichi il recupero di base imponibile, possibilmente senza appesantire la burocrazia fiscale sulle imprese e i cittadini. Ad ogni modo, l'aspettativa di recuperare evasione fiscale per 6,6 miliardi appare ottimistica, considerato che per recuperare 5,6 miliardi di entrate è stato necessario un provvedimento straordinario, come lo scudo fiscale per il rimpatrio dei capitali. In conclusione, siamo di fronte a una manovra correttiva dura, ma necessaria, che ha un impatto recessivo, che si sarebbe potuto mitigare con alcuni miglioramenti nella selezione dei tagli e nelle misure di accompagnamento per gli investimenti delle imprese. Una manovra che affida la ripresa dell'economia e in parte lo stesso riequilibrio della finanza pubblica al tiraggio della domanda estera, stimolata dal deprezzamento dell'euro, e alla benevolenza della Banca centrale europea. è un atto di grande responsabilità politica e nel superiore interesse del Paese approvarla senza indugi. Chiedo Signor Presidente, la manovra finanziaria in discussione nasce da esigenze che possono anche ritenersi condivisibili per il riequilìbrio dei conti. Ciò non significa che essa non debba essere dettata a principi di equità e giustizia. Essa deve rappresentare un momento fondamentale per delineare e dare concretezza a provvedimenti di cui si avverte la necessità anche per migliorare lo Stato sociale, il benessere dei cittadini, ma soprattutto per eliminare quelle anomalie che non sono degne di un Paese civile ove vige la democrazia. È il momento in cui vengono definite le priorità, soprattutto basandosi sul contesto sociale attuale. Vorrei inoltre soffermarmi su una grave carenza di questa manovra che mi sta particolarmente a cuore evidenziare: non si affronta il tema delle invalidità in forma sistemica. La disabilità è materia complessa ed occorre affrontarla innanzi tutto su due presupposti, cioè la coscienza civica e l'impatto sociale. Mi viene da pensare che occorra sovvertire l'attuale punto di osservazione: comunemente si tende a pensare che la disabilità sia un peso per la società; io sostengo che sia più logico pensare che allo stato attuale è la nostra società che si pone come un peso per il disabile, proprio perché la questione deve essere posta in un'ottica diversa. Si consideri quanto sia difficile l'inserimento nel mondo del lavoro o l'essere accantonato da parte da una società che non riconosce al disabile gli stessi diritti o almeno le stesse aspettative di qualsiasi cittadino. Infatti, al disabile viene riconosciuta una pensione da fame, che certamente mina la dignità della persona ed è scandalosa per un Paese civile ed evoluto. Meno male che si è evitato, con un'inaspettata illuminazione sulla via di Damasco degli estensori del disegno di legge, che si procedesse ad una sciagurata revisione delle percentuali per accedere al diritto. la dimostrazione che si conosce ben poco il mondo della disabilità e che neanche esiste una cultura sociale per trovare soluzioni organiche ed efficaci per favorire l'inserimento a pieno titolo nella nostra società. Mi preme sottolineare in questo contesto che poco viene destinato al mondo della disabilità, il quale anzi viene mortificato con i tagli agli enti locali, dalle Regioni ai Comuni.

Cito solo poche parole: «I loro diritti sono diritti di tutte le persone. Nei territori più efficienti si è sviluppato un sistema di servizi integrati per assicurare alle persone con disabilità i livelli essenziali di diagnosi, cura, riabilitazione». In realtà, credo altro punto critico riguarda il blocco del *turnover* nel settore della sanità. Le risorse umane sono altamente qualificate ed ogni figura professionale svolge un ruolo determinante. Inoltre, sono gravi le carenze in talune specialità mediche. Per fare un riferimento ancora più stringente, mi richiamo alla difficile situazione organica del personale infermieristico, tecnico e di assistenza alla persona. Da alcuni anni le aziende sanitarie fanno ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, anche a personale straniero, proprio per rispondere alle più immediate esigenze. Ricordo, tra l'altro, che nella sanità le prestazioni vengono erogate 24 ore al giorno. Pertanto, in carenza di personale di personale l'unico rimedio può essere la chiusura di reparti ospedalieri o la riduzione di prestazioni territoriali. Inoltre, la dirigenza delle aziende sanitarie ha già obiettivi di spesa che le Regioni hanno imposto e quindi era già previsto un eventuale taglio nell'utilizzo delle risorse umane. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, ossia la necessità di cui alla manovra di ridurre i costi, il recupero delle risorse può avvenire mediante provvedimenti attuativi di norme di equità fiscale, sebbene ci sia da considerare che il mancato rispetto degli standard dei livelli essenziali di assistenza provoca costi sociali di molto superiori a quelli che vogliono essere gli ipotetici risparmi.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sette mesi fa in quest'Aula si discuteva il disegno di legge finanziaria per il 2010. In quell'occasione, diversi esponenti della maggioranza affermavano che il nostro Paese, che aveva retto meglio degli altri all'impatto della crisi, avrebbe dovuto affrontare nei mesi successivi una sfida per il futuro: quella di ritrovare una capacità di crescita, nonostante le condizioni di finanza pubblica. Veniva ribadita la necessità di trovare uno spunto e uno spirito riformatore. Intenzioni e parole apprezzabili, alle quali purtroppo non sono seguiti i fatti, visto che oggi ci troviamo a discutere di un provvedimento che si contraddistingue per la totale assenza di crescita, nonché per il suo carattere iniquo e complessivamente molto debole in termini di efficacia. Non vi è alcuna indicazione sulla strategia da seguire per favorire il recupero di competitività del nostro Paese nel contesto internazionale, una competitività oggi già debole ed ulteriormente deteriorata da questi tagli indiscriminati alla spesa, che colpiscono molto poco gli sprechi e le inefficienze, mentre tagliano i diritti dei lavoratori, delle piccole imprese, degli studenti universitari e, in generale, di tutti i cittadini. In particolare, peseranno sulla crescita i tagli ai trasferimenti alle Regioni, alle Province e ai Comuni, strangolati da questa manovra, ma soprattutto peseranno quelli che agiscono su alcuni capitoli del bilancio dello Stato: mi riferisco ai tagli al settore dei lavori pubblici, ove le riduzioni delle dotazioni delle missioni di spesa dei Ministeri intervengono, in particolare, sul diritto alla mobilità e sulla missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», aggiungendosi ai numerosi interventi già realizzati in sede di approvazione della finanziaria. Non è possibile che non riusciate a capire, cari colleghi della maggioranza, che la qualità del sistema delle reti infrastrutturali strategiche - sia materiali che immateriali è uno dei fattori cruciali dello sviluppo e della crescita di ogni Paese: esso incide in modo determinante sui costi della produzione di beni e servizi, sulla competitività delle imprese, sul loro accesso ai mercati e sugli scambi commerciali. È un fattore cruciale anche per la qualità della vita e per la coesione sociale: dalla qualità delle reti infrastrutturali e dei servizi di rete dipende la mobilità delle persone, la fruizione di beni essenziali (l'acqua, l'energia elettrica, il gas), le relazioni interpersonali (il telefono, le poste), la diffusione delle informazioni e delle conoscenze (Internet), il monitoraggio dei fattori di rischio ambientale e sociale ed una crescente parte dei servizi socio-sanitari. Vi pare poco? Se ho deciso di soffermarmi su questo punto è perché credo che la regolazione, lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali siano tra i problemi e tra le sfide fondamentali che gli Stati contemporanei devono affrontare. Ciò vale, ovviamente, anche per l'Italia. Se lo sviluppo delle infrastrutture è un indice dello stato di salute di un Paese e della sua capacità di governo, il modo in cui questa manovra ha affrontato il tema è invece l'esempio lampante di un Esecutivo allo sbando, in cui l'assenza di una capacità di governo ha portato a misure che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo. Basti pensare che in questo decreto, che avrebbe dovuto avere tutt'altra finalità, ha trovato posto anche la riforma della Conferenza dei servizi. La finalità di un tale intervento dovrebbe essere quella di rendere più spedita l'approvazione di tutti i progetti che necessitano del via libera di più enti pubblici, a partire quindi proprio dalle opere infrastrutturali ed energetiche. In realtà, l'obiettivo di questa norma è solo quello di annientare il ruolo delle amministrazioni preposte alla cura di interessi che voi ritenete "oppositivi" e che a noi invece preme proteggere, ossia quelli attinenti alla tutela dei valori e dei beni giuridici di rilevanza costituzionale quali la salute, il paesaggio, la difesa del suolo e delle risorse naturali, la promozione culturale, l'ambiente.

strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale. Tutto ciò Tutto ciò non solo è in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, non solo dimostra che non siete a conoscenza del fatto che la VAS e la VIA sono due procedure distinte, perché incidono su ambiti diversi (la VAS su piani e programmi, la VIA su progetti e opere), ma soprattutto smentisce quello che, solo qualche giorno fa, avevate sottoposto alle Commissioni parlamentari:

specificando che essa costituisce un procedimento autonomo. E allora questo cos'è? È l'ennesimo refuso che avete dimenticato di correggere? Sarebbero queste le misure capaci di sbloccare il Paese? Sarebbe questo partire lancia in resta contro una normativa di tutela ambientale il rimedio all'immobilismo del Paese? Ma questo è solo il primo esempio di questa vostra cieca modalità di procedere, preoccupata solo di buttare dentro tale testo il maggior numero possibile di interventi, smentendo le finalità iniziali e dimenticando anche stavolta che esiste un Parlamento - siamo qui, basta guardarsi intorno - e che su certe scelte occorrerebbe confrontarsi. Invece, voi avete recepito in Commissione, con un tris di emendamenti, il contenuto dell'accordo per l'autotrasporto siglato il 17 giugno scorso sul tavolo del Ministero; avete praticamente esautorato il ruolo della 8ª Commissione, ne avete ne avete vanificato il lavoro ed avete condiviso un accordo che non è stato firmato da tutti i rappresentanti del settore, che apporta notevoli innovazioni e che non risolve i nodi strutturali della questione. Persino Confindustria, a voi tanto cara, si è detta contraria a questo accordo. In un contesto in cui le risorse per la realizzazione delle autostrade sono al minimo (anche quelle per completare i lotti della Salerno-Reggio Calabria) e le risorse per le ferrovie sono prese quasi solo dalle Regioni (e riguardano solo le carrozze), tutto quello che avete saputo fare con questa manovra è stato limitarvi a prevedere il sostegno finanziario di alcuni interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, attraverso il recupero di risorse che non vanno a gravare direttamente sulle finanze pubbliche. La scelta di revocare i mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2006 libera al massimo 635 milioni, destinati in via prioritaria al finanziamento del MOSE e per la restante parte alla prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche (praticamente briciole). Durante la «notte dei miracoli» - quella quella di venerdì sera - in Commissione bilancio è stato approvato l'emendamento «salva filobus» che, anziché togliere i finanziamenti là dove non sono stati aggiudicati i contratti di appalto, li toglie solo se non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte o delle richieste di invito previste dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori. Così gli 86 milioni destinati ai filobus veronesi sono salvi. Questo significa che, quando si vuole, si può. Non vi sono purtroppo in questo provvedimento cenni al blocco delle cosiddette grandi opere e, in particolare, al blocco di un'opera controversa e molto costosa (e, aggiungerei, del tutto inutile): il ponte sullo Stretto di Messina, il cui costo è stimato attualmente in 6,3 miliardi di euro, gran parte dei quali a carico diretto dello Stato o di organi al cento per cento controllati dallo Stato (quali l'ANAS o le Ferrovie). Nonostante quasi nessun progresso dei lavori sia stato realizzato, mentre si continuano a pagare i lauti stipendi della società di gestione, la realizzazione del ponte non viene minimamente intaccata, lasciando che l'operazione di pulizia si concentri sulle infrastrutture finanziate e non ancora trasformatesi in cantiere. La parte pubblica di investimento per il ponte ammonta ad almeno 2,5 miliardi, anche se alcune delle cifre sono ancora riservate. Ma, se avesse ragione la Corte dei conti a dubitare che il traffico privato sarà sufficiente a coprire il resto dei costi, è facile prevedere oneri ulteriori a carico dello Stato. Badate bene, l'intera manovra è volta a recuperare 25 miliardi di euro. Cancellare l'impegno del ponte di Messina sarebbe equivalente a circa un quarto dell'intera operazione. Avete deciso poi di rinnovare, tramite gara, la concessione dell'autostrada del Brennero. Tale concessione doveva scadere nel 2005; a quella data, l'autostrada era stata interamente ammortizzata. Gli azionisti, che negli anni Settanta avevano investito una cifra quasi simbolica (meno di 3 miliardi di vecchie lire), si ritrovavano in cassa circa 600 milioni di euro di euro di liquidità e titoli, a fronte di un patrimonio contabile di 287 milioni di euro e di «un fondo ferrovia» di 302 milioni di euro.

la società ha avuto un margine operativo lordo di 138 milioni di euro e un utile netto di 66 milioni di euro. perché dovrebbe essere riassegnata nuovamente la concessione, visto che l'autostrada è da tempo giunta a compimento e il nuovo concessionario avrebbe solo due compiti: esazione dei pedaggi e manutenzione. Lo Stato, tramite l'ANAS, avrebbe potuto appaltare ciascuno dei due ruoli a imprese private, considerando anche che la pluralità di potenziali concorrenti produrrebbe effetti economici notevoli, e incamerare tutto il ricavo netto dell'autostrada. Si sarebbero evitati così i costi, le incertezze e le insidie di gare per concessioni di lunga durata, nonché eliminati i gravosi costi amministrativi di società che hanno per solo oggetto la gestione di un tratto di autostrada. Tali spunti inducono a una riflessione importante su tale manovra. Invece no: la vostra linea e rimasta la stessa del 2005, prevedendo che l'ANAS pubblicherà un bando di gara per l'affidamento di una nuova concessione entro settembre; che il bando dovrà indicare il valore della concessione e le modalità di pagamento; che il subentrante dovrà continuare gli accantonamenti al «fondo ferrovia». Nodo, quello del «fondo ferrovia», rimasto negli anni anomalo

prevedere la continuità del finanziamento al tunnel del Brennero, e stabilire che gli introiti per il tunnel potranno essere usati da parte del concessionario per realizzare opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento (da Modena a Bolzano), opere che potranno essere anche urbane o consistenti in gallerie. Si è data così una robusta spinta anche alla realizzazione del traforo delle Torricelle. Insomma, Verona ormai la fa da padrona. Nel 2005, insieme alla decisione di rinnovare la concessione per l'autostrada del Brennero, era stata tentata anche l'istituzione di nuovi pedaggi autostradali. «Squadra che vince non si cambia» e quindi, oltre che il nuovo bando di gara per l'autostrada del Brennero, coerentemente con le linee del 2005, dal 1° luglio, come sapete, sono scattati anche i pedaggi sui raccordi autostradali e sulle autostrade gestite direttamente dall'ANAS, a cui tra l'altro, si somma anche un'altra intuizione geniale che avete avuto: quella dell'aumento del canone per tutta la rete autostradale in concessione, di cui dirò a breve. Il risultato è un euro di sovrappedaggio per autovetture e moto e 2 euro per i veicoli pesanti su 26 caselli di concessionarie autostradali interconnessi a raccordi e autostrade dell'ANAS. Il sistema - come si dice sempre - è provvisorio, e resterà in vigore solo fino alla fine del 2011, quando il sistema di pedaggiamento entrerà a regime su 22 arterie ANAS, tra cui potrebbero esserci il raccordo anulare di Roma, la Roma-Fiumicino e la Salerno-Reggio Calabria. La misura dovrebbe fruttare 83 milioni nel 2010, 200 milioni nel 2011 e 315 milioni da quando andrà a regime: tutti soldi che consentiranno allo Stato di risparmiare sui trasferimenti all'ANAS per investimenti e manutenzioni straordinarie. Occorre rilevare, però, che il sistema di pedaggiamento a regime va costruito e, soprattutto, vanno costruiti i caselli; il tutto entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2012, salve le solite proroghe. Nell'immediato, quindi, gli oneri per rendere esigibile il pedaggiamento probabilmente saranno maggiori dei benefici, con il risultato che tutto questo ha un costo che pesa interamente sui cittadini tutti, in particolare sui pendolari che ogni giorno sono costretti a spostarsi sulle arterie di collegamento con le grandi città. Stiamo parlando di quegli stessi pendolari a cui voi state tagliando anche i treni e gli autobus, costringendoli così ad usare l'auto, a pagare di più e ad inquinare il doppio. Scaricando sulle Regioni e sugli enti locali la maggior parte dei tagli e cancellando i trasferimenti statali, si distruggerà in sostanza il trasporto pubblico locale, con effetti devastanti sulle risorse destinate ai bus, metro e ferrovie locali ed inevitabili conseguenze per milioni di pendolari e studenti, gravissimi disagi e nuovi disservizi. Il ministro Matteoli purtroppo persevera nell'errore di negare l'evidenza dei 3,5 miliardi di euro di tagli e delle conseguenze che ne deriveranno a partire dalla seconda metà del 2010 e nel 2011, smentendo gli stessi governatori regionali che da più di un mese denunciano l'irresponsabilità di tali scelte. Questa scure che sta per abbattersi sugli enti locali non colpirà, però, tutti allo stesso modo. La Lombardia, il Lazio, la Puglia e la Campania in particolare soffriranno una diminuzione pesantissima, con fondi bloccati e rinnovamento del parco macchine rinviato *sine die*. Sorte migliore non toccherà alla Toscana. Dal Fondo trasporti della Regione Lombardia spariranno 314 milioni: stiamo parlando di cifre importanti.

della maggioranza abbiate smarrito anche quel minimo di buon senso che vi restava. Non è così che si ripara agli errori commessi e, soprattutto, tutto ciò non può essere fatto sempre pesare sulle spalle dei cittadini. Basta tornare alla questione dell'aumento dei prezzi che graveranno sugli automobilisti, per avere una chiara dimostrazione di quanto detto: sommando il sovrapprezzo del pedaggio con l'incremento del canone che le concessionarie dovranno corrispondere all'ANAS si arriva ad un aumento, in alcuni tratti, pari al 18-20 L'aumento dei canoni che le concessionarie autostradali dovranno pagare all'ANAS sarebbe stata una misura anche condivisibile, considerati i continui benefìci di cui le stesse godono. Peccato che le concessionarie hanno già inventato una sorta «clausola di prevenzione», mirata a rendere innocui gli effetti. La protezione consiste proprio nella possibilità automatica di rivalersi sulle tariffe. Lo schema che si delinea è pressoché il seguente: l'automobilista paga, le concessionarie riscuotono, l'ANAS incassa. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vi aveva invitato a riesaminare le normative vigenti in materia di regolazione. Anziché contribuire alla diminuzione delle tariffe voi le avete aumentate. Non è forse questa una delle tante inefficienze a cui ci avete abituato? Questo modo di governare il Paese non è forse responsabile delle «lacrime e sangue» che verseranno gli italiani? Io credo che la risposta sia sì, ma è più comodo usare uno dei tanti scudi che a voi piacciono tanto. E stavolta lo scudo è l'Europa.

«Signor Presidente, è sotto gli occhi di tutti, in questi giorni, la vicenda che riguarda la cosiddetta inchiesta sull'eolico. Si tratta di fatti i cui aspetti penali sono di stretta competenza della magistratura della quale il Parlamento ha il dovere di difendere l'autonomia. Il Gruppo del PD vuole affrontare la questione politica che deriva da fatti che coinvolgono i vertici del principale partito del nostro Paese, esponenti di governo e magistrati. La questione è di tale rilevanza che riteniamo urgente che il Parlamento ne possa discutere con serietà e profondità. Dopo le inchieste sulla Protezione civile, dopo le dimissioni del ministro Scajola e dopo le dimissioni del ministro Brancher, emerge un quadro inquietante nel quale agiscono, fianco a fianco, importanti rappresentanti della politica e delle istituzioni e personaggi che hanno avuto ruolo in vicende molto gravi e molto serie della storia repubblicana e che oggi esercitano funzioni di consiglieri, esecutori, suggeritori e hanno potere di condizionamento in merito a scelte proprie di organi e poteri pubblici. La invitiamo pertanto a chiedere al Presidente dei Consiglio, a nome delle senatrici e dei senatori del PD, di presenziare a un dibattito parlamentare sulle condizioni della nostra Repubblica, sulle responsabilità politiche, sulle misure che il Governo intende assumere per contenere la gravità di quanto continua a emergere. L'onorevole Berlusconi non è mai venuto nell'Aula di Palazzo Madama se non in occasione dell'insediamento del suo Esecutivo. Crediamo che un dibattito di tale rilevanza richieda, oggi, la sua presenza.

rispetto al comparto delle politiche ambientali questa manovra ha effetti pesanti, per quello che dice e molto anche per quello che non dice. Passo sopra ai tagli lineari che colpiscono il Ministero dell'ambiente come gli altri Ministeri. Sono comunque tagli importanti: oltre 30 milioni di euro in meno per ognuno dei prossimi tre anni. Ma il comma 24 dell'articolo 7 nasconde una mannaia ben più pesante: il dimezzamento - lo ripeto: il dimezzamento - dei fondi per gli enti gestori dei parchi nazionali. In Italia ci sono oggi 23 parchi nazionali,

dal 2011 i fondi per i nostri parchi nazionali crollerebbero a 24 milioni di euro, il che vuol dire più o meno 17 euro per ogni ettaro di area protetta, esattamente un terzo della media di quanto i Paesi europei spendono per i loro parchi parchi nazionali. L'impatto di questa misura sui parchi nazionali italiani sarebbe non solo drammatico, ma in molti casi esiziale, perché le risorse a disposizione degli enti parco scenderebbero spesso al di sotto della soglia necessaria a pagare gli stipendi e le bollette. Sostanzialmente si metterebbe in discussione l'esistenza stessa di questi organismi, che sono pezzi dello Stato e della pubblica amministrazione e che non sono enti o fondazioni private, anche se forse, dietro questa misura, c'è l'aspirazione a farli diventare tali. Si sta parlando, è bene ricordarlo, di alcuni dei maggiori tesori naturalistici e ambientali non solo d'Italia, ma del mondo: dal parco d'Abruzzo, allo Stelvio, al Circeo, al Gargano, alle Cinque terre. che dà lavoro, diretto o indiretto, a quasi 100.000 persone e che si rivolge ad un pubblico di 30 milioni di visitatori ogni anno. Mi soffermo poi su due articoli specifici della manovra: uno è l'articolo 19, che riguarda la cosiddetta regolarizzazione delle case fantasma, l'altro l'articolo 45, sui certificati verdi. Per quanto riguarda l'articolo 19, la maggioranza e il Governo hanno ripetuto più di una volta che non si tratta di un condono edilizio mascherato e nemmeno della premessa per un nuovo condono edilizio. Poi però, pochi giorni fa, su «Il Sole 24 ORE» di domenica scorsa, non un passante, ma il ministro Calderoli ha dichiarato che, grazie a questa misura, i Comuni italiani potranno recuperare 5 miliardi di euro, per cento del valore - stimato in 50.000 euro a immobile - dei due milioni di immobili fantasma. Ora, poiché più di metà di questo patrimonio è costituito da immobili abusivi interamente o parzialmente , delle due l'una: o la parte abusiva di questo patrimonio resta illegale, e allora l'incasso per i Comuni sarà molto meno della metà di quanto stimato dal ministro Calderoli, oppure questa parte abusiva del patrimonio delle case fantasma verrà sanata, e allora si tratterà - né più né meno - di un condono. Sull'articolo 45 in queste settimane si e scritto molto e molte sono state le prese di posizione, anche di rappresentanze del mondo produttivo, a cominciare da Confindustria, che ne ha chiesto la soppressione. Sostanzialmente questa è una misura che cancella l'obbligo per il GSE, il gestore della rete elettrica, di ritirare i titoli di produzione delle fonti rinnovabili che il mercato non assorbe; si sta parlando di una forma di incentivo allo sviluppo delle fonti rinnovabili. Tra l'altro, faccio presente rispetto a quanto ha detto prima di me la presidente Finocchiaro, che un sistema certo e stabile di incentivi alle energie rinnovabili è anche uno dei principali mezzi di difesa dalle speculazioni e dagli abusi che pare stiano emergendo proprio in questi giorni da alcune inchieste giudiziarie. Bene, se questa misura fosse rimasta così come'era prevista all'inizio, la manovra finanziaria avrebbe messo in ginocchio un settore industriale molto vitale e promettente del nostro Paese. Una prima modifica proposta dal relatore eliminava, tra l'altro, l'unico argomento plausibile che si può utilizzare a sostegno di questo articolo 45 che non porta un euro in più nelle casse del fisco ma che, si diceva, consentirà di alleggerire le bollette elettriche di circa 600 milioni di euro. Bene, una prima modifica proposta dal senatore Azzollini eliminava anche il risparmio per gli utenti (questi 600 milioni), prevedendo di utilizzarli per un fondo per la ricerca: in pratica, lo trasformava in una nuova tassa. Nella versione attuale, con un gioco di prestigio degno della finanza creativa della stagione d'oro del ministro Tremonti, rimane la tassa alimentata dai vecchi incentivi CIP6, che restano in bolletta ma che vengono utilizzati per fare cassa, scompare il risparmio per gli utenti e si riduce, a partire dal 2011, l'importo a disposizione del GSE per il ritiro dei certificati in eccedenza, dilazionando così, ma certo non azzerando, l'incertezza per tutti gli operatori. Faccio presente che l'Italia, entro il 2020, in base al pacchetto clima che il nostro Paese e questo Governo hanno deciso di sottoscrivere pochi mesi fa, deve raddoppiare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

il mancato rifinanziamento del credito di imposta del 55 per cento alle ristrutturazioni energetiche degli edifici. Questa era un misura, introdotta a suo tempo dal Governo Prodi, che aveva dato grandi risultati (aveva fatto aprire decine e decine di migliaia

degli interessi del fisco. Ecco, credo che più di tante scelte sbagliate, questa scelta che non c'è nella manovra finanziaria proposta dal Governo dia la misura di quanto il Governo e la maggioranza sappiano solo, e spesso male, rincorrere i problemi e le emergenze senza avere la minima idea di quale possa o debba essere il futuro del nostro Paese.*(Applausi *(LNP)*. Signor Presidente, colleghi senatori, credo sia sicuramente evidente in questo periodo che l'aspetto socio-economico che maggiormente caratterizza il nostro tempo è la crescita delle interdipendenze tra i Paesi e quindi tra i diversi sistemi economici e sociali che compongono il nostro pianeta. È la cosiddetta globalizzazione, il cui incedere ha ormai sicuramente il mondo in un'unica grande area nella quale i fenomeni più diversi riescono a diffondersi con una rapidità e un'intensità che nei casi di crisi sono tali da poter creare effetti devastanti. Ma questo credo ormai lo abbiamo capito tutti, perché ne stiamo subendo gli effetti. In questo senso, la recente speculazione sull'euro, andandosi a saldare sulla parte finale della crisi economica, rischiava di produrre effetti gravemente destabilizzanti che era ed è necessario prevenire attraverso una serie di contromisure strutturali impostate in riferimento ad un orizzonte di largo periodo e di ampie vedute. Riteniamo che la manovra su cui siamo chiamati ad esprimerci risponda sicuramente appieno alla necessità di far fronte alle difficoltà poste dall'evoluzione del quadro economico e, soprattutto, che abbia in sé i contenuti per garantire la stabilizzazione finanziaria e incentivare la competitività economica. La manovra, proprio perché strutturale e di carattere generale, incide in profondità sul nostro sistema economico che è, di fatto, interessato in ogni sua componente, inclusa anche l'agricoltura. Il richiamo al settore agricolo è utile in riferimento a due aspetti che, sebbene non siano granché rilevanti rispetto ai grandi numeri economici della manovra, sono tuttavia da ritenere significativi per i loro contenuti impliciti. Mi riferisco, in particolar modo, alle disposizioni inerenti l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) ed a quelle relative al programma dei termini per il pagamento delle multe pregresse, le cosiddette quote latte. l'ENSE è inserito nella lista degli enti pubblici da chiudere. Nell'operare in tal senso si è evidentemente omesso di considerare che l'ENSE non riceve contributi pubblici, che si autofinanzia attraverso lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e che, addirittura, reinveste gli avanzi di gestione a beneficio del settore delle sementi. Credo sia particolarmente significativo segnalare che l'ENSE ha, tra gli altri, il compito di certificare le sementi, ossia di svolgere una funzione che, oltre ad essere di assoluta importanza ai fini della tracciabilità e della sicurezza alimentare, è necessaria al fine di garantire il rispetto delle norme che regolano la produzione di sementi; tant'è vero che in ogni Paese dell'Unione europea sono presenti strutture analoghe al nostro Ente nazionale delle sementi elette. Ciò è di notevole importanza, soprattutto in un momento importante come questo in cui sembra che gli OGM, tutte le colture OGM, stiano prendendo il sopravvento non tanto nel gradimento dei consumatori, della gente, ma in una parte della politica che piano piano, in maniera strisciante, credo inizi a promuovere gli organismi geneticamente modificati. Noi della Lega Nord invece siamo di parere contrario. La Lega Nord ritiene che occorra salvaguardare valori quali la certezza della genuinità del prodotto, l'identità, la tradizione, la qualità dei prodotti agricoli dei nostri territori. Dobbiamo preservare la sana agricoltura tramandataci dai nostri padri. In questo senso, ritengo degno di attenzione il caso dell'ENSE che, pur nell'ambito di una manovra complessa e dei grandi numeri, è stato, comunque, posto all'attenzione nel corso del presente passaggio parlamentare. Credo che particolare attenzione debba essere rivolta anche alle decisioni assunte in materia di quote latte. Su questo argomento ritengo indispensabile operare alcune precisazioni in quanto, come spesso accade, questa materia si presta alle peggiori speculazioni e strumentalizzazioni politiche. Si è detto, in questi giorni, che le norme introdotte in Commissione tutelano quei pochi che, volontariamente, si sono posti fuori dal sistema. Lo stesso ministro Galan ha dichiarato ieri da Bruxelles che in quest'Aula parlamentare, in questo ramo del Parlamento «viene difeso un piccolo manipolo di trasgressori». dal fatto che nessuno pensa che ben oltre la metà del latte che beviamo non è prodotto nelle nostre stalle, ma viene importato dall'estero a prezzi stracciati e prodotto chissà come come e chissà dove. Mentre noi impediamo ai nostri allevatori di produrre, permettiamo al latte straniero di essere commercializzato nei nostri negozi. Un latte che, peraltro, spesso e volentieri è confezionato con la dicitura a dir poco ingannevole: «prodotto e confezionato in Italia». A tal proposito, credo sia giusto, doveroso ed eticamente corretto, ricordare e sollecitare al ministro Galan la legge sull'etichettatura, sul *made in Italy* alimentare, approvata dal Senato circa 5 mesi fa, ma ferma alla Camera. La sua approvazione porterebbe un grosso beneficio al valore del latte dei nostri agricoltori e, sicuramente, aumenterebbe il reddito di tutto il settore agricolo del nostro Paese. Dispiace esprimersi in questi termini, ma quanto sta accadendo è talmente paradossale da apparire grottesco. Con la proroga dei pagamenti a fine 2010, stiamo solo cercando di dare un po' di respiro economico ai nostri contadini,

questo punto, e io credo che debba riflettere anche il Ministro dell'agricoltura con tutto il Governo. Chiaramente, invitiamo a un lavoro più forte, ad andare in Europa e a ricontrattare ulteriormente la nostra parte di quote latte, così come hanno fatto con successo i suoi predecessori, soprattutto il ministro Zaia, che un anno fa riuscì ad ottenere ben il 6 per cento di quote in più per i nostri allevatori. Il problema vero, la genesi di tutto, com'è stato detto parecchie volte in quest'Aula parlamentare, sono state le trattative fallimentari condotte in Europa 25 anni fa dall'allora ministro Pandolfi. Trattative disastrose, largamente penalizzanti per i nostri agricoltori. Oggi stiamo lavorando per rimediare agli errori del passato. Le norme introdotte in Commissione prevedono, infatti, una semplice proroga delle scadenze da applicarsi non, come stato detto recentemente, ad «un manipolo di trasgressori», a tutti i soggetti interessati all'unico fine di dare respiro ad un settore che sta patendo sicuramente come gli altri, e forse più di altri, gli effetti della crisi, proprio perché gravato dal peso delle multe pregresse. Una norma, quindi, pienamente coerente con lo spirito del presente decreto legge che - giova credo a tutti ricordarlo - non persegue solo l'obiettivo della stabilizzazione finanziaria, ma anche quello del recupero della competitività competitività che, nel settore del latte, si sta cercando di favorire con le norme in questione. In considerazione degli effettivi contenuti delle norme e delle reazioni sproporzionate che le stesse hanno suscitato, viene da pensare che quanto sta accadendo non sia tanto finalizzato al ritiro della proroga, bensì ad innalzare un fuoco di sbarramento verso altre e più significative iniziative che, in materia di quote latte, sarà necessario assumere sicuramente al di fuori del presente decreto. Ci riferiamo in particolare alle recentissime sentenze del TAR del Lazio, che hanno ribadito l'incongruenza tra la normativa europea e le norme nazionali sulle compensazioni prioritarie e, quindi, hanno di fatto dichiarato l'illegittimità delle multe comminate tra il 1995 e il 1996 e il 2001 e il 2002, ossia delle multe che i nostri allevatori hanno pagato e stanno continuando a pagare. ci riferiamo anche ai risultati delle indagini condotte dai Carabinieri che, così come accadde una quindicina di anni orsono con la cosiddetta commissione Lecca, hanno evidenziato la presenza di gravi anomalie che inficiano i dati produttivi e che, di conseguenza, gettano ombre sulla legittimità delle multe imposte ai nostri allevatori. Il settore lattiero-caseario è una componente di assoluta importanza del nostro sistema agro-alimentare, il cui valore si estende oltre il settore agricolo, andando a interessare il complesso delle attività economiche che, con esso, hanno rapporti sul territorio. Per questo motivo riteniamo che sia funzionale, non all'interesse di un manipolo di trasgressori, ma all'interesse dell'intera comunità nazionale, evitare che una componente del nostro sistema socio-economico sia portata al fallimento per circostanze, come le multe sulle quote latte, la cui legittimità è continuamente messa in discussione non da soggetti di parte ma da organi di Stato, come accade oggi con il TAR del Lazio, con i Carabinieri o come spesso è accaduto, in passato, con altri tribunali o con commissioni di indagine costituite per legge, nonché presiedute da importanti esponenti della Guardia di finanza. Ciò abbiamo tenuto ad evidenziare affinché le questioni inerenti alle norme in materia di quote latte proposte del presente decreto non siano strumentalmente mischiate con ben più gravi problemi di fondo che dovranno essere affrontati sicuramente in altre sedi. Da un lato, dunque, la proroga delle scadenze per il pagamento delle multe che, in coerenza con gli obiettivi del presente decreto, è una norma unicamente finalizzata a dare ristoro finanziario alle imprese già provate dalla crisi; dall'altro, e in dall'altro, e in altra sede, la risoluzione del problema della legittimità delle multe pregresse e, quindi, della restituzione della certezza del diritto ad un settore il cui futuro sviluppo è funzionale

Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, entro subito nel merito delle cose per dire che questa finanziaria non risponde alle esigenze reali del Paese. A ben guardare tra la miriade di tagli e soppressioni, il Governo, ancora una volta, non affronta alcun nodo strutturale, anzi, se ce ne fosse ancora bisogno, sancisce la differenza di velocità tra il Nord e il Sud dell'Italia. Il risanamento delle finanze viene sempre presentato come il risultato di interventi contabili, dunque di esclusiva natura tecnica, ma alla fine dei conti ci sono sempre settori risparmiati ed altri più colpiti dalla scure dei tagli. Il dato di partenza, a mio avviso, è il record mai toccato prima dal debito pubblico: oltre 1.812 miliardi di euro. Gli incassi del fisco calano: secondo i dati contenuti nel bollettino delle entrate tributarie diffuso dal Dipartimento delle politiche fiscali, nei primi quattro mesi del 2010 le entrate tributarie sono state pari a 108,8 miliardi di euro,

che dichiara che il dato sul debito «non preoccupa, è inerziale. E la manovra è fatta proprio per questa inerzialità». Proprio il settore del pubblico impiego, con particolare riferimento alla scuola, è tra le vittime principali di questa manovra, insieme alle Regioni, agli enti locali e alla spesa farmaceutica. E poi c'è il grande sconfìtto, cari colleghi, il Mezzogiorno, che scivola sempre di più verso le Regioni più povere dell'Europa, mentre il Nord, grazie all'attenzione costante della Lega di Bossi, che anche stavolta ha dettato patti e condizioni ai soci di Governo, può confrontarsi con le risorse industriali del Nord Europa. Leggendo il testo della manovra, mi sono chiesto che fine abbia fatto il federalismo fiscale. Se ne parla tanto, per diciassette giorni abbiamo avuto anche un Ministro delegato all'applicazione del federalismo, poi scomparso. Tremonti ha presentato con il consueto ottimismo l'introduzione delle zone a burocrazia zero per il Meridione, in deroga alla normativa in vigore che poteva essere corretta senza introdurre per forza un nuovo provvedimento. Il Ministro ci ha spiegato che servirà ad agevolare l'apertura delle piccole e medie imprese, ma io credo che le piccole e medie imprese avrebbero bisogno di misure che ne agevolino la crescita, capaci di renderle competitive, per radicarsi nei territori e strutturare la loro attività. E le aziende medio grandi? Nella manovra finanziaria se ne parla timidamente, quasi che in Italia non ce ne fosse più bisogno, quasi che potessero bastare solo le piccole e medie imprese. Non mi pare superfluo sottolineare che anche questa misura finirà col penalizzare il Sud. Esattamente come i tagli alle Regioni, agli enti locali e agli enti e istituti culturali e di ricerca di cui si è disposta la soppressione. La mannaia cade in maniera indiscriminata, e invece bisognava razionalizzare valutando le situazioni e tenendo presenti, nel caso degli enti cancellati, quali sono davvero inutili. Quando si chiede, come ho fatto io con alcuni colleghi - anche della maggioranza - di salvare il Centro studi di Portici o di «saldare il debito» con l'Istituto degli studi filosofici di Napoli, non si interviene per campanilismo, ma per non sottrarre al territorio - e Dio sa quanto Napoli, la Campania e il Mezzogiorno ne abbiano bisogno - presìdi importanti di crescita, veri e propri motori di sviluppo culturale, intellettuale, civico. Ancora una volta questo Governo, come è già accaduto per la gestione della crisi dei rifiuti in Campania, interviene senza un disegno organico e la sensazione è che il risparmio a colpi d'accetta non si tradurrà in guadagno, cioè in reali entrate per le casse dello Stato. Su tutto, a fronte di mortificazioni vere e proprie inflitte alla scuola e alla sanità, regna sovrana una grande confusione. Come faranno, chiedo al ministro Tremonti, le Regioni e gli altri enti territoriali a gestire le riduzioni così considerevoli previste dal Governo? Un taglio così drastico riduce lo spazio di autonomia di questi enti, che al Sud in modo particolare è già molto esiguo, lasciando il territorio ancora più esposto all'avanzata della criminalità organizzata, che invece le risorse le ha e non esita ad utilizzarle, dando la scalata ai mercati per aumentare i propri capitali. Questo è uno dei miei più grandi timori ed è una questione prioritaria da affrontare se realmente si vuole far uscire il Sud dall'isolamento in cui mafia, camorra e 'ndrangheta lo stanno progressivamente costringendo. Ritengo che il Governo avrebbe dovuto esprimersi in maniera molto più netta per sbarrare il passo alla criminalità, organizzata.

ed è bene che si cominci, ma non sono convinto che la strada scelta dal Governo sia efficace. Come dimenticare il maxicondono dello scudo fiscale e il rischio che ad avvantaggiarsene, ancora una volta, sia la criminalità organizzata? per il Mezzogiorno, si sbandiera la fiscalità di vantaggio, ma non si capisce come potrà essere attuata se dall'altro lato si tagliano risorse importanti e aiuti di Stato. Per non parlare del cosiddetto regime fiscale di attrazione europea, chiaramente anticostituzionale e in contrasto con le norme comunitarie. Al di là degli spot e della Al di là degli spot e della facile propaganda, a farne le spese sono i giovani, che devono fare i conti - è il caso di dirlo - con il blocco delle assunzioni e delle carriere nel pubblico impiego e con i tagli dei contratti a tempo determinato. Mancano il senso dello Stato e il senso della comunità, per cui altro che equità e solidarietà! Sono un illusorio e inutile miraggio di giustizia civile e sociale. Tutto ciò a rischio il futuro di tante giovani generazioni del nostro Paese e la vita stessa della democrazia; altro che crescita e sviluppo! Credo che questo Governo e questa maggioranza si debbano far carico di questa tragedia, di questo discredito che le istituzioni del Paese vivono, per tentare di recuperare una stagione di speranza e di futuro, specialmente per le aree più deboli del Paese.

la situazione di difficoltà economica, finanziaria, occupazionale e di competitività rende necessaria e scontata l'emanazione di una manovra correttiva dei conti pubblici. Tutti i Paesi europei sono intervenuti per reagire alla crisi internazionale in maniera anche più consistente dell'Italia, ma soprattutto in maniera più strutturale. La manovra che stiamo discutendo si fonda su due grandi pilastri fondamentali: riduzione di costi e semplificazione nella pubblica amministrazione e nella politica; lotta all'evasione. Le misure previste per la correzione dei conti pubblici con scelte precise di ridimensionamento della spesa pubblica sono in gran parte condivisibili,

con abolizione di innumerevoli enti inutili, accorpamenti di strutture e servizi, passaggi di competenze e responsabilità a Regioni, Province e Comuni; inoltre, si sarebbe potuto preparare concretamente la via del federalismo fiscale. Faccio un esempio: dopo tutte le lamentele delle Regioni per i tagli previsti in questa manovra e l'amara convinzione che lo Stato centrale non riuscirà mai a far emergere e ottenere l'iscrizione regolare nel catasto delle case e delle unità immobiliari in generale ed eventuali relativi contratti d'affitto, perché non cogliere le cogliere le proposte avanzate e lungamente discusse in Commissione di trasferire le competenze in merito alle Regioni e agli enti locali, lasciando loro le entrate tributarie, creando un'imposta sostitutiva unica sugli immobili, e la cedolare secca sugli affitti, affidando loro la gestione e i controlli? Questa proposta è stata ripresa dal Governo nella relazione al Parlamento sull'attuazione del federalismo fiscale come misura da adottare in futuro. Perché allora non attuarla concretamente in questa manovra dando un segnale concreto di un intervento strutturale di decentramento, di semplificazione, di lotta all'evasione fiscale e di intervento a favore dei cittadini? Signor Presidente, questa è un'occasione persa per passare dalla politica degli annunci alla politica dei fatti concreti. Si sente tanto in questa manovra la mancanza di un profilo strutturale e di un incentivo allo sviluppo economico. Il Governo in Commissione bilancio ha sempre fatto riferimento all'Europa e alla necessità di adeguamento anche da parte dell'Italia. Condivido la necessità ed il concetto, ma soltanto se si creano i presupposti di partenza adeguati. Nelle misure previdenziali della manovra il Governo ha inserito l'innalzamento a 65 anni dell'età pensionabile delle donne nella pubblica amministrazione. Una misura di adeguamento a quelle vigenti negli altri Paesi europei,

È ora di realizzare una seria politica della famiglia e di seguire proprio in questa materia l'Europa. Il Governo non può fare riferimento all'Europa solo quando gli conviene. Un altro esempio è il continuo riferimento alla necessità di adeguamento all'Europa in campo fiscale. Anche in questo caso il semplice raffronto generalizzato non rispecchia una politica fiscale approfondita e seria. Siamo i primi in Europa per il prelievo fiscale sul lavoro e quindi nella classifica dei contribuenti più tassati con obblighi burocratici insostenibili. Le piccole e medie imprese stanno soffocando sotto i continui aumenti di obblighi burocratici e di difficoltà finanziarie quasi insormontabili e non vedono prospettive future. La nostra politica fiscale attuale è molto lontana da quella dei Paesi europei che vorremmo prendere a modello. Iniziamo con l'adeguamento della tassazione vigente, abbassando le aliquote alla media europea così da far rifiatare imprese e contribuenti e concentriamoci su un sistema di controlli seri e mirati, equamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, per combattere l'evasione fiscale. Evitiamo di aumentare o reintrodurre obblighi burocratici esagerati a scapito di tutti i contribuenti, punendo come al solito i contribuenti onesti; ma introduciamo tecniche nuove come quelle adottate in altri Paesi europei, che hanno dato ottimi risultati. Per quanto riguarda il contributo al Patto di stabilità interno per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano previsto all'articolo 14, ricordo al Governo e specialmente al ministro dell'economia e che le province di Trento e Bolzano hanno nel novembre 2009 firmato l'accordo previsto nell'articolo 27 della legge delega sul federalismo fiscale.

e la partecipazione delle stesse al conseguimento degli obiettivi di perequazione, di solidarietà e del Patto di stabilità interno. Pertanto, devo precisare che noi già per primi abbiamo contribuito alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e mantenuto gli impegni assunti con la firma dell'accordo siglato. Ci aspettiamo che anche il Governo rispetti gli accordi raggiunti. La delicatezza del momento richiede misure più credibili una riforma della politica fiscale, il cui obiettivo principale sia la ripresa economica del Paese attraverso misure che non si limitino ad aggiungere oneri fiscali, previdenziali e burocratici a carico dei contribuenti.

stato difficilissimo in uno stato di incertezza e di chiusura da parte del Governo, mai visto fino ad ora. Signor Presidente, per fare una politica che risponda ai problemi dei cittadini e alle esigenze del Paese nel rispetto delle norme europee ci vorrebbe un confronto parlamentare più aperto, interventi strutturali, più disponibilità al dialogo da parte del Governo e più scelte condivise in Parlamento.

i nuovi, ennesimi, tagli alle forze dell'ordine. In essi ben si riassumono le caratteristiche dell'intero decreto, dall'accanimento con cui vengono limate fino all'osso le risorse già scarse delle fasce più deboli della popolazione, all'ottusità con cui si penalizzano settori chiave per lo sviluppo ed il benessere dell'intera società, a cominciare - appunto - dal comparto sicurezza. Rincuora sapere che in un recente sondaggio le forze dell'ordine risultano l'istituzione più apprezzata nel Paese: 1'83 per cento degli italiani intervistati ha espresso molta o moltissima fiducia nei loro confronti. Per quanto tempo ancora - viene da chiedersi, manovra alla mano - continuerà ad essere così? Per quanto ancora gli uomini e le donne che indossano la divisa potranno continuare a svolgere degnamente il proprio lavoro? Già oggi - come noto dalle numerose proteste sindacali si va avanti con enormi sacrifici. Tra i primi atti di questo Governo (la manovra d'estate 2008 per il triennio 2009-2011), abbiamo registrato riduzioni al Ministero dell'interno pari ad oltre 1 miliardo e mezzo di euro nel complesso. Nelle finanziarie e nei provvedimenti successivi si è proseguito sulla stessa linea: tagli, sospensione degli straordinari, stop alla manutenzione e alle riparazioni dei veicoli e «Siamo figli di tutte le opposizioni e orfani di tutti i Governi» hanno denunziato più volte gli agenti di Polizia. Ed è vero. La situazione era già grave durante la scorsa legislatura, anche il precedente Governo - non ho difficoltà ad ammetterlo - ha proceduto a consistenti tagli nei confronti del comparto sicurezza. Eppure, è solo negli ultimi due anni che, oltre al danno, le forze dell'ordine hanno conosciuto la beffa:

della futura maggioranza, quando l'attuale *Premier* in persona assicurò: «Noi non taglieremo mai, mai, mai alle forze di polizia; la sicurezza è priorità della nostra agenda politica». solo parole. La sicurezza sul territorio non è oggi in alcun modo migliorata. È solo diminuito il tempo che le televisioni padronali dedicano a questo tema. Il Governo continuamente sbandiera i successi raggiunti nella lotta alla criminalità organizzata, ma voglio ricordare che quei successi, spesso frutto di indagini avviate da tempo, sono da ascriversi unicamente all'abilità e alla perseveranza di magistratura e forze dell'ordine: nessun ministro, di destra o di sinistra, può prendersene il merito. In ogni caso, nulla o poco hanno a che fare con la sicurezza sul territorio, ossia con la piccola e media criminalità, che quotidianamente affligge e preoccupa la gente. Sono certo che la maggioranza non ignora queste fondamentali distinzioni; eppure continua sulla strada di sempre, quella delle beffe (dalle ronde ai militari in strada) e quella dei tagli. Con l'attuale manovra, la Polizia porta a casa un taglio di quasi 560 milioni di euro, un colpo attutito ben poco dall'emendamento del Governo che *in extremis* ha restituito ai comparti sicurezza e difesa 160 milioni per il biennio 2011-2012, ossia 40 milioni l'anno ciascuno. È facile il calcolo: si tratta di 12 euro al mese per ciascun dipendente dei due comparti, irrisoria per coprire tutti gli scatti di carriera, obiettivo per il quale il fondo è stato istituito. Al comparto sicurezza e difesa, nel complesso, vengono sottratti oltre 1,6 miliardi di oltre alle retribuzioni ferme al 2010, al blocco negli avanzamenti stipendiali, ai notturni, straordinari e festivi non pagati e alle liquidazioni rateizzate; senza contare il balletto sulle tredicesime che, al di là della sua conclusione, ha rappresentato l'ennesima mortificazione per tutti i dipendenti pubblici minacciati da questa misura. Cos'è tutto questo se non «mettere le mani nelle tasche degli italiani»? Nessuno tra le fila dell'opposizione, onorevoli colleghi, vuole nascondersi dietro un dito. Sappiamo bene che la crisi esiste e che a tutti sono richiesti dei sacrifici. Per amore di verità, tuttavia, vorremmo che questa situazione la si ammettesse chiaramente dai palazzi del Governo e dai banchi della maggioranza e, allo stesso tempo, vorremmo che questi sacrifici fossero imposti seguendo la logica del buon senso e della solidarietà sociale: non ai più deboli, dunque, e non a settori vitali come la sicurezza, la ricerca e la sanità. Mi sia consentita, infine, una riflessione. Sappiano le forze dell'ordine quanto sia inutile questo mio intervento, al pari degli interventi precedenti e di quelli che seguiranno. È triste e preoccupante constatare ancora una volta l'inutilità assoluta del lavoro dell'Aula, in un contesto nel quale, da questa parte dell'emiciclo, si rimane sempre, irrevocabilmente, inascoltati, e dall'altra parte - la vostra parte, onorevoli colleghi della maggioranza - si è condannati alla totale obbedienza a direttive calate dall'alto. Stiamo parlando di manovra finanziaria, una manovra che ha interessato tutto il Paese:

è che - come peraltro già avvenuto negli anni 2008 e 2009 - il Governo ha inteso affrontare i temi centrali della finanza pubblica in una misura anticipata, ricorrendo ad un provvedimento che di fatto anticipa i contenuti e le misure della futura legge di stabilità - già legge finanziaria - prima della pausa estiva. Questa decisione, dettata dall'emergere a livello internazionale di una turbolenza sui mercati finanziari ben lungi dall'essere esaurita, ha il vantaggio di permettere una tempestiva definizione delle misure che, in buona parte, scatteranno dal 2011, consentendo nei prossimi mesi una messa a punto nel dettaglio delle misure oggi anticipate ed individuate. Occorre d'altro canto sottolineare come la presente manovra, proprio perché dettata dall'urgenza di rassicurare i mercati internazionali in ordine all'andamento del *deficit* e del debito pubblico del prossimo triennio, non costituisce una riforma compiuta, anche se sono presenti alcuni elementi strutturali che cercherò di evidenziare. C'è però, innanzitutto, l'urgenza di mettere in sicurezza i conti dello Stato per evitare che attacchi speculativi mettano in seria difficoltà il meccanismo di collocamento del debito pubblico. È dunque una situazione molto delicata, vista la rilevanza dell'indebitamento statale; ma l'Italia si trova, forse per la prima volta, in condizioni migliori di altri Paesi europei che, non a caso, oggi sono costretti a manovre anche più pesanti, come accade addirittura in Germania. Infatti, tutte le rilevazioni statistiche avallate dagli osservatori internazionali confermano che, per quanto riguarda i contraccolpi

o la Gran Bretagna, dove l'indebitamento delle famiglie e la crisi del mercato immobiliare stanno determinando situazioni preoccupanti. Inoltre, per quanto attiene alle finanze pubbliche, anche la situazione del *deficit* attuale è migliore di quella di altri Paesi, come ad esempio Francia e Germania, tale da richiedere una manovra di dimensioni meno ampie. All'Italia e al ministro Tremonti è stato tributato in sede europea un riconoscimento unanime per l'efficacia delle misure assunte sul piano Anche le recenti innovazioni introdotte per interpretare il Patto di stabilità europeo, considerando il livello di indebitamento del sistema Paese alla luce della somma del debito pubblico e privato, mette l'Italia in una condizione relativa decisamente migliore che non nel passato più o meno recente. Occorre tuttavia prendere realisticamente atto che la crisi economica scoppiata nel 2008, e con conseguenze che la fanno paragonare a quella del 1929, ha richiesto alle finanze pubbliche degli Stati di tutto il mondo uno sforzo tale da determinare un aumento rilevante del debito pubblico, ribaltando la tendenza al contenimento che era stata imposta dalla costruzione della moneta unica. C'è da dire che proprio la lezione del '29 ha insegnato agli Stati ad agire con forme di aiuto massicce in via anticipata, prima del pericoloso avvitamento della crisi, rinviando ai momenti successivi la gestione delle conseguenze inevitabili che ciò avrebbe avuto sui debiti pubblici. Sugli Stati, che sono dovuti intervenire per evitare il collasso dell'economia mondiale, pesa dunque l'aumento degli aggregati monetari che è stato necessario immettere sul mercato per operare il salvataggio del sistema. Secondo i dati più recenti, la massa monetaria è cresciuta negli anni più recenti nei principali Paesi sviluppati o emergenti in modo vertiginoso, passando da un indice statistico pari a 100 nel 2005, a 130 per gli Stati Uniti (nel 2010), 137 nell'area Euro, 149 per i Paesi europei dell'OCSE e 227 per la Cina (ma forse il ragionamento sulla Cina va valutato diversamente, perché ha crescite diverse). Si tratta di una molla carica al massimo, pronta a far schizzare in alto l'inflazione quando le condizioni della ripresa economica mondiale ne provocheranno il rilascio. Ma la soluzione inflazionistica per erodere il debito pubblico cumulato in funzione anticrisi presenta delle controindicazioni da non sottovalutare. Dal punto di vista economico, ha senso fintanto che l'ammontare complessivo del debito è sostanzialmente inferiore al PIL. La manovra però diventa meno efficace man mano che il debito cresce fino a superare il 100 per cento del PIL, perché in questo caso il costo dei maggiori oneri per interessi finisce con l'eliminare il beneficio della riduzione in termini reali del debito. Dal momento che, Italia a parte (in cui il rapporto tra debito e PIL è ben superiore all'unità), diversi Paesi europei si stanno avvicinando rapidamente a questa soglia, tale possibilità appare oggi quasi completamente depotenziata. La stabilità della moneta europea dipende dunque da una strategia complessa di intervento, che rifugge da ogni scorciatoia e da ogni soluzione unilaterale (quali alcuni interventi che la Germania ha voluto adottare sul sistema sul sistema borsistico, che peraltro forse avevano una natura più interna che esterna). In primo luogo, occorre che i singoli Stati, come stanno in effetti facendo, pongano in atto politiche di rigore volte a ridurre la spesa pubblica, tagliando in particolare quella improduttiva, per ridurre il *deficit* e mettere a disposizione risorse per lo sviluppo. Infatti, la strategia di riduzione del peso del debito non può che passare da un aumento della capacità di crescita dell'economia europea, che oggi viene sfidata dalle economie emergenti, perché il rapporto debito-PIL può essere ridotto sia agendo sul numeratore sia agendo sul denominatore (quindi è fondamentale aumentare la capacità di crescita). In secondo luogo, occorre intaccare la spesa pubblica improduttiva, fenomeno particolarmente evidente in un Paese come l'Italia, in cui lo Stato intermedia ben oltre la metà del prodotto interno lordo. Di fatto, la manovra predisposta dal Governo per la prima volta punta per due terzi sul contenimento della spesa e solo per un terzo sull'aumento delle entrate, principalmente mediante il recupero dell'evasione fiscale (stimata ben oltre i 100 miliardi di euro). L'impianto sostanziale del decreto-legge n. 78 del 2010 punta dunque su due pilastri fondamentali: razionalizzazione delle spese pubbliche e lotta all'evasione fiscale. Nell'ottica dell'eliminazione degli sprechi anche potenziali, il legislatore ha inteso guardare non solo in prospettiva futura, ma addirittura al passato, più esattamente a tutte quelle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti, evidentemente già decisi sulla base di altre leggi finanziarie, non sono stati utilizzati. In tal caso, occorre ricordare che, sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato, le autorizzazioni di spesa per gli anni 2007, 2008, 2009 sono state definanziate, cioè depurate del vincolo a quell'obiettivo per cui erano state stanziate. L'operazione non coinvolge solo ciò che l'amministrazione, per motivazioni varie, non ha utilizzato, ma anche quanto di quegli importi non è stato impiegato: si prevede, infatti, che il residuo di quegli stanziamenti, riallocato alla voce «entrata» del bilancio dello Stato, sarà riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli statali. Le finalità del suddetto decreto-legge (stabilizzazione finanziaria e competitività economica), perseguite con una manovra che richiederà evidenti sacrifici al Paese, sono accompagnate anche da riforme strutturali, ovvero non contingenti e legate alle emergenze contabili, quale quella del sistema pensionistico, imposta certamente dall'Unione europea, ma con effetti di lungo periodo sul nostro Paese. Appare opportuno sottolineare come

operando nell'emergenza, l'eventuale mancata differenziazione su base meritocratica potrebbe rischiare di frustrare le aspettative dell'apparato statale. Il secondo pilastro della manovra consiste invece nelle entrate che deriveranno dal contrasto all'evasione. La lotta all'evasione fiscale, oltre che un dovere morale, rappresenta un utile strumento per la diminuzione della pressione fiscale. Una parte consistente delle nuove entrate discenderà dunque dall'accelerazione delle procedure di riscossione (su questo si è agito anche in sede di Commissione), nonché dalla partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento.

utili correttivi, pur tenendo invariata l'entità dei saldi della manovra. Soprattutto, ci si è concentrati raccogliendo le indicazioni provenienti dal sistema pubblico e da tutti gli interlocutori delle realtà sociali ed economiche ed intervenendo con le correzioni consentite.

è decisamente negativo. Le soluzioni proposte dal Governo sono inadeguate, sia per far fronte alla grave situazione in cui versa la spesa pubblica, il *deficit* ammonta infatti a 82 miliardi di euro secondo le stime del 2010, la manovra si rivela inadeguata per rilanciare l'economia ed il lavoro, per affrontare le vere emergenze sociali quali il fenomeno della disoccupazione, della riduzione dei redditi ed anche i bassi consumi che contraddistinguono la nostra società e la nostra economia. Come hanno scritto 100 economisti italiani in una lettera aperta al Governo - credo che le loro parole siano da ascoltare, da leggere e da considerare di riflessione - la crisi mondiale, esplosa nel 2008, è tuttora in corso e non essendo intervenuti sulle cause strutturali, di fatto non ne siamo mai usciti. Il Governo ha cercato di limitare i danni della crisi, a scapito delle fasce più deboli della popolazione, ma sembra aver dimenticato che sono proprio i cittadini comuni i principali attori economici, sia in termini di singoli che di nuclei familiari. Da cosa deriva il nostro giudizio negativo su questa manovra? Voglio ricordare un dato: questa manovra voleva addirittura colpire le persone disabili. Alla fine, la fine, la maggioranza ha capito che quello era proprio un errore gravissimo. Non si sarebbero eliminati i falsi invalidi in quel modo. Sull'eliminare i falsi invalidi, se di falsi invalidi si può parlare nel nostro Paese,

Certo, un intervento sui conti pubblici è necessario, ma questa soluzione di politica economica va integrata con misure che permettano alle famiglie e alle imprese di attutire gli effetti che tali sacrifici porteranno sui redditi. Accertata l'inutilità degli interventi *una tantum*, servono invece scelte precise, circoscritte e misurabili. Le risorse che potrebbero arrivare dalla lotta all'evasione fiscale devono servire per abbassare l'imposizione fiscale, per garantire i redditi delle famiglie e dei lavoratori e non per altro. La manovra, per come è stata scritta, non solo trascura la dimensione familiare per i nuclei esistenti, ma evita ancora una volta di affrontare il tema della forte denatalità che colpisce l'Italia da almeno 20 anni. È fondamentale partire dalle famiglie per far ripartire l'Italia. Servono delle scelte indicizzate che consentano di valutare gli interventi in base al reale costo della vita. Questa manovra invece non è una scelta: è una non scelta, è, in fondo, anche una negazione dell'esistenza della famiglia come nucleo sociale fondamentale, non solo e non tanto riconosciuto dalla Costituzione. Dal momento in cui è stata scritta la Costituzione ad oggi, la famiglia ha subìto delle radicali e profondissime trasformazioni, però era e continua a rimanere fortunatamente l'elemento pulsante e centrale della nostra società. Quindi, credo che avremmo dovuto, grazie anche a questa manovra, cercare di proteggere e difendere il nostro vero valore aggiunto, che è la famiglia. Non possiamo far finta di non vedere che il nostro Paese soffre di un grave *deficit* demografico. È qui che la politica deve dimostrare di essere credibile, con interventi mirati a sostegno della natalità, e più vicina alle giovani famiglie che devono scegliere con serenità figli. Rispetto alla Francia siamo di fronte ad un suicidio demografico. La parola è eloquente per dimostrare la situazione. Questo Paese non dà speranza e non ha futuro

di coniugare l'altra importante scelta per le donne: mettere a frutto le loro risorse professionali in campo lavorativo. Queste tre scelte si possono coniugare:

c'è bisogno di individuare alcune priorità su cui lavorare. Chiediamo dei sacrifici ad alcuni per far entrare maggiori risorse nelle casse dello Stato, ma al tempo stesso dobbiamo essere in grado di individuare alcune priorità. Ciò che questo Governo non sta facendo è proprio tale individuazione. Il Governo toglie ai poveri e lascia ai ricchi: lasciatemi usare una frase forse

È come se voi snobbaste la politica familiare, considerando la famiglia come un freno al mercato invece che una forza propulsiva all'interno della società:

Concludendo, ritengo che il Governo abbia perso un'importante occasione per offrire al Paese un assetto fiscale e finanziario più stabile, per aiutare imprese e famiglie, per attuare una reale lotta all'evasione fiscale e per realizzare interventi a sostegno della crescita e dell'occupazione. Come ricordava Adam Smith, il padre dell'economia moderna, la società non può sussistere tra coloro che sono sempre pronti a danneggiarsi e a farsi torto l'un l'altro. Ancora una volta voglio ricordare qui le parole di un grande filosofo rinascimentale, Francesco Guicciardini, che forse ci offre la soluzione a questi problemi, all'incapacità che questo Governo ha dimostrato con questa manovra.

dall'esigenza, avvertita a livello internazionale, di placare le pressioni negative dei mercati finanziari e quindi per evitare all'Italia il rischio Grecia. Così, in attuazione di un comune intento espresso in sede europea, anche il nostro sistema finanziario ha dovuto adeguarsi ad un meccanismo di stabilizzazione monetaria. Questo però non vuol dire che il decreto-legge al nostro esame non fosse necessario. Al contrario, è stato spesso definito un'opportunità che il nostro sistema Paese attendeva da tempo, considerando soprattutto l'alto livello di indebitamento pubblico.

una congiuntura economica da tempo condizionata da fattori negativi, con la finalità implicita di rimettere in moto il meccanismo dello sviluppo. La crisi ha indebolito la stessa moneta europea, e questo perché la necessità di salvare molte banche in crisi ha appesantito lo *stock* del debito pubblico

ma l'Italia è anch'essa esposta alle incertezze che caratterizzano il sistema finanziario internazionale e per questo motivo ha dovuto varare una manovra finanziaria, come stanno facendo gli altri Paesi europei grandi e piccoli.

La manovra, dunque, nel biennio avrà effetti finanziari strutturali per complessivi 24 miliardi di euro. Obiettivo degli interventi è ricondurre il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2012 al di sotto del 3 come previsto dal Trattato di Maastricht. Le misure sono incentrate su tagli alla spesa pubblica, sulla riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione. Dal lato delle entrate, le misure si concentrano sul contrasto all'evasione fiscale e contributiva. Viene decisa la partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione, a fronte di un maggiore introito sulle somme recuperate. Sono rafforzate le verifiche incrociate fra INPS e Agenzia delle entrate; viene introdotta la tracciabilità attraverso le fatture telematiche, mentre sono escluse nuove imposte o aumenti di quelle esistenti. linee generali, ma è chiaro che il testo varato inizialmente dal Governo è stato sostanziosamente modificato in Commissione bilancio. Va detto poi in termini molto positivi dall'esame preliminare in Commissione è scaturito un testo della manovra che ha impegnato maggioranza ed opposizione in un confronto che potremmo definire esemplare e del quale devo ringraziare il presidente Azzollini. Evidentemente, l'approfondito dibattito parlamentare ha dovuto affrontare una rotta turbolenta tra contenimento della spesa pubblica e la ricerca difficile, ma necessaria, di un criterio di assoluta equità sociale, con una oculata ripartizione degli oneri sociali.

e che ci auguriamo possa invece trovare presto una soluzione positiva e rassicurante. Trattandosi però di aperta conflittualità tra istituzioni della Repubblica, è indispensabile trovare un punto d'incontro, perché il rischio è quello di contraddire lo stesso impegno programmatico ed elettorale della maggioranza a favore del federalismo. il taglio dei servizi ai cittadini potrebbe risultare un *boomerang* per la stessa maggioranza. Intervenire in modo indiscriminato penalizzando le Regioni sarebbe palesemente contraddittorio. E intervenire favorendo le Regioni cosiddette virtuose può sembrare politicamente legittimo, ma risulterebbe un modo sicuramente discriminatorio di concepire il federalismo, che è la grande riforma istituzionale che dobbiamo realizzare in questa legislatura. Ma veniamo ad alcuni aspetti specifici della manovra. La manovra interviene in modo incisivo sulla spesa corrente. È però necessario, a mio giudizio, attuare anche misure che incentivino i consumi, perché alla contrazione dei consumi consegue un necessario ridimensionamento dell'offerta. Rispetto all'andamento del ciclo economico, la manovra si colloca nella fase di consolidamento della ripresa, ma bisogna tener presente che la crisi del biennio 2008-2009 non ha ancora esaurito i suoi effetti sia sull'economia reale sia sulla finanza pubblica.

- è stato sostenuto anche il rischio che potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi in futuro, qualora si presentasse uno scenario diverso e ancora più sfavorevole di quello assunto alla base della manovra in esame. Mi voglio poi soffermare su una delle misure che ha fatto più discutere e che ha riguardato l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne. Dopo la sentenze di condanna per il nostro Paese da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea si è aperto il dibattito, si sono confrontate le tesi, si sono cercate Il pensionamento anticipato delle donne è stato da sempre giustificato come risarcimento per il lavoro che esse svolgono in famiglia durante la vita. Ma questo risarcimento, in realtà, perpetua lo stesso circolo vizioso che vorrebbe eliminare. Infatti, l'ammontare della pensione in Italia viene calcolato in rapporto ai contributi versati durante il periodo lavorativo; quindi, la minore partecipazione al mondo del lavoro e la minore retribuzione portano le donne ad avere una pensione più povera rispetto a quella degli uomini in un periodo della vita in cui, invece, si rendono necessarie maggiori risorse. È importante allora ciò che è previsto nell'emendamento presentato dal relatore e dalla Commissione, che fa confluire le maggiori entrate che derivano dall'equiparazione dell'età pensionabile nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per interventi dedicati a politiche sociali e familiari e all'esigenza di conciliare lavoro e vita familiare. È infatti imprescindibile che le risorse ottenute dall'innalzamento dell'età pensionabile devono essere, come *conditio sine qua non*, destinate alle donne proprio per conciliare lavoro e famiglia. allora che se si vuole ottenere l'effetto di incoraggiare e dare impulso al mercato del lavoro, così che più donne possano trovare occupazione, è necessario utilizzare anche la leva fiscale. Per questo ho presentato un emendamento, poi accolto come ordine del giorno dal Governo e dal relatore, che impegna il Governo a destinare una quota di questo Fondo strategico ad interventi legislativi diretti ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia a favore delle donne che lavorano. Sono convinta, infatti, che per favorire una partecipazione quantitativamente e qualitativamente più elevata delle donne al lavoro sia necessario configurare strumenti di politica fiscale specifica che aumentino la disponibilità economica e finanziaria delle lavoratrici che, in questo modo, saranno loro a scegliere quali servizi siano più adatti alle proprie esigenze. Vorrei, inoltre, ricordare l'ordine Vorrei, inoltre, ricordare l'ordine del giorno sull'educazione finanziaria, che ritengo molto importante, presentato ed accolto all'unanimità dalla Commissione e dal Governo: un punto importante e più volte richiamato nelle relazioni del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, e del presidente della CONSOB, Lamberto Cardia,

svolgevano le Casse di risparmio e le Banche del Monte insieme all'esercizio del credito. Le fondazioni, dunque, rappresentano una risorsa fondamentale da tutelare per sostenere lo sviluppo sociale, culturale, politico ed economico del nostro Paese. È stata introdotta non soltanto la possibilità di elevare la percentuale di possesso dei beni immobiliari delle fondazioni dal 10 al 15 per cento, ma è stata anche introdotta la previsione che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'economia ora e l'Autorità che sarà istituita poi presentino una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle dalle fondazioni. Sono contraria al ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza e al conseguente voto di fiducia. Per questo motivo voglio oggi ringraziare il relatore che ha condotto magistralmente i lavori in Commissione, dando ampio spazio agli interventi dei senatori

essa si è trasformata in un'opportunità positiva, innanzitutto per il contenimento della spesa, come era nostro dovere nei confronti dell'Europa, e secondariamente per l'attuazione di un criterio di assoluta equità.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, da settimane il Governo dice al Paese che la manovra finanziaria che stiamo discutendo è una manovra voluta dall'Europa, che richiede agli Stati membri un riequilibrio dei loro conti pubblici per contrastare la crisi, le pressioni speculative, per difendere l'euro e sostenere la ripresa. Conveniamo tutti di essere di fronte a una situazione seria, molto seria, e che c'è bisogno di una manovra pesante per mettere in ordine i conti pubblici. Ma in Europa ci sono scenari economici e sociali diversi. Il nostro Paese in questi ultimi terribili anni ha visto crescere il proprio debito pubblico, peggiorare sensibilmente il rapporto *deficit-*PIL, non ha registrato sostanziali miglioramenti nel proprio sistema strutturale e infrastrutturale e soffre di un'endemica ed elevatissima evasione fiscale e contributiva, che grava tanto sui lavoratori quanto sulla parte sana e produttiva del Paese. Il Paese è ancora in piedi, non tanto per gli esiti di un'accorta politica del Governo, ma soprattutto grazie alla propria vocazione al risparmio Il Paese è ancora in piedi grazie alla creatività e alle capacità imprenditoriali e di lavoro di quella parte produttiva responsabile che sopravvive pagando tutte le inefficienze del sistema. In questi due anni il Governo ha sbagliato la lettura della crisi, arrivando persino a negarla, e ha sottovalutato le conseguenze, risultando totalmente inabile a creare un rinnovato quadro di sostegno alla ripresa. Non ha condotto un'efficace lotta all'evasione fiscale, non ha avviato un processo organico di semplificazione e razionalizzazione del sistema Paese, ha lasciato sole le piccole imprese. Di fatto, anche questa manovra si caratterizza per l'assenza di qualsiasi misura destinata direttamente al sostegno e allo sviluppo dell'economia. Non ci sono interventi o idee in grado di sostenere le famiglie e il sistema produttivo italiano. Non ci sono misure per il sostegno della domanda e dell'offerta. Solo tagli per ben 25 miliardi di euro, la maggior parte dei quali agli enti locali e, di conseguenza, alla parte più debole della popolazione per quanto riguarda servizi, sanità, scuola e formazione professionale. Si pensa di mandare in pensione le donne a 65 anni senza pensare a misure, a strumenti seri, solidi ed efficaci di sostegno al *welfare*. Nella manovra ci sono tagli, riduzioni di spesa che influiranno pesantemente nel prossimo triennio sulle imprese a causa del taglio lineare del 10 per cento degli stanziamenti di bilancio, taglio che non fa distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale. Ma sappiamo tutti che in un periodo di crisi non si possono tagliare gli investimenti perché sono essenziali per il rilancio dell'economia. Le piccole e medie imprese, prive di adeguate risorse finanziarie e di credito, saranno ancora le più esposte alla concorrenza sempre più aggressiva dei nuovi attori dell'economia emergente. Solo nella missione «competitività e sviluppo delle imprese» assistiamo a tagli di 216 milioni di euro negli anni 2011 e 2012, altri 94 nella missione «energia e diversificazione delle fonti energetiche». Per quanto riguarda il turismo, i tagli lineari sottraggono ulteriori 11 milioni dopo i pesanti tagli già operati con le finanziarie 2009 e 2010. Quindi per il turismo - consentitemi l'espressione - stessa spiaggia, stesso mare: vale a dire niente di niente. Le proposte del Partito Democratico non accolte dal Governo prevedevano agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio alberghiero, estendendo agli imprenditori turistici turistici le agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio; agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici; la riduzione dell'aliquota IVA sui pacchetti turistici rivolti al turismo sociale o per migliorare l'erogazione dei buoni vacanza. Un intervento concreto, ben diverso da quello di dubbio gusto pensato dal ministro Brambilla e dal Presidente del Consiglio, che ha prestato la propria voce a uno spot di carattere autarchico che sprona gli italiani italiani a rimanere in Italia, anziché pensare di portare un numero sempre maggiore di turisti stranieri. Sembra che il ministro Brambilla ed il presidente Berlusconi non si rendano conto che se la gente non va in vacanza non è per ignoranza o indifferenza verso le bellezze nazionali, ma perché non

Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, siamo davanti ad una manovra che prova a mantenere - come questa mattina chiara ed eloquente ha detto il presidente Azzollini - gli impegni presi con l'Europa e a contrastare una crisi finanziaria che ha avuto manifestazioni clamorose in Paesi a noi vicini come la Grecia. Mettere in sicurezza i nostri conti pubblici, tenere a bada il nostro debito pubblico e la sua incidenza in termini di costo e ancor di più di rischio, rallentare un *trend* di crescita della spesa pubblica che in questo ultimo decennio è cresciuta ad un ritmo del 4,5 per cento (più di quattro volte la crescita della ricchezza nazionale) mi sembra siano stati i fattori decisivi della scelta del Governo di intervenire con tempestività per correggere i conti ed allinearli agli impegni di stabilità assunti in Europa. Si è detto da più parti che questa manovra è non solo necessaria, ma per tanti versi sostenibile rispetto alle scelte fatte in altri Paesi europei, e con caratteri di equità. Del resto, basta guardare a quanto accaduto in Francia dove, per contenere un deficit dell'8,2 per cento e riportarlo al 3,2 per cento nel 2012, si è varata una manovra di 100 miliardi di euro, di cui la metà è rappresentata da tagli di spesa pubblica. Per non dire della Germania della Merkel, con un manovra quadriennale di 80 miliardi di euro attraverso aumenti di imposte e tagli di spese.

L'Inghilterra di Cameron si accinge da gennaio ad aumentare l'IVA dal 17,5 al 20 per cento e ad incrementare la tassa sulle rendite finanziarie dal 18 al 28 con una manovra da 80 miliardi di euro che prevede il taglio di 400.000 posti pubblici ed il congelamento delle retribuzioni.

Questo è il contesto in cui si muove la manovra italiana, che prova a sollecitare un contenimento della spesa attraverso meccanismi che spingono alla sua razionalizzazione e qualificazione, lanciando una sfida che è morale prima che politica a tutti i centri di spesa e a tutti gli attori che intervengono nella formazione della spesa pubblica.

anch'essa importante e dall'alto valore morale - che consiste nel rafforzamento delle azioni di contrasto al gravissimo ed ormai insopportabile, per l'intera comunità nazionale, fenomeno dell'elusione e dell'evasione fiscale. Credo che tutti dobbiamo apprezzare questa assunzione di coraggio da parte del Governo, che non rinuncia ad affrontare due questioni strutturali della politica del nostro Paese (e non da oggi), che sono appunto rappresentate dall'incontenibile partito della spesa, che ha portato la spesa pubblica a raddoppiarsi in un decennio da 450 miliardi di euro a più di 800 miliardi di euro, e dalla questione fiscale, che tiene insieme livelli di evasione stimati in oltre 100 miliardi annui miliardi annui di mancato gettito ed una pressione fiscale che si è trasformata in oppressione, con livelli che superano il 42 per cento di tassazione sui redditi. una contraddizione - peso e costo degli apparati ed alta pressione fiscale - che esige risposte chiare e segnali non ambigui, su cui il Governo si sta muovendo con una determinazione che va apprezzata nella lotta agli sprechi, nel dimagrimento degli enti e delle burocrazie centrali, regionali e locali: in una parola, nell'affievolimento del peso degli apparati e del loro costo. ciò sta avvenendo nella semplificazione delle procedure per i cittadini e per le imprese, poggiando sulla responsabilizzazione degli stessi e sui controlli *ex post*. In questa direzione, signora Presidente, sono da salutare con fiducia sia l'idea delle zone a burocrazia zero nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno che le misure per introdurre elementi di fiscalità di vantaggio da negoziare al più presto con l'Europa, volendo confermare che alle necessarie politiche di rigore si devono inevitabilmente accompagnare politiche di sviluppo azionando le leve della semplificazione e dei vantaggi fiscali per costruire fattori di attrazione proprio nelle aree a ritardo di sviluppo. una manovra rigorosa per lo sforzo di razionalizzazione della spesa pubblica ed equa per la lotta che si accinge a rilanciare al fenomeno della evasione

ha generato elementi distorsivi nelle dinamiche dello sviluppo e spesso l'inutile impiego di ingenti risorse pubbliche senza esiti per l'attecchimento di processi di accrescimento delle reti produttive e di evoluzione dei sistemi economici e sociali. modo, sono segnali qualificanti le misure tese a premiare il rientro dei ricercatori con incentivi fiscali per docenti e ricercatori che tornano in Italia e le misure che premiano la produttività nel settore privato con sgravi fiscali e contributivi per il 2011. Si è molto discusso sul peso e sul contributo che le Regioni e gli enti locali sono chiamati ad offrire a questa manovra e ai suoi saldi, che mi sembra non siano discussi. Spero ed auspico che il livello di cooperazione e di dialogo si possa recuperare anche a valle di questa approvazione, tutti consapevoli che il Paese intero è di fronte a sfide non più rinviabili che portano il nome di una verifica della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli. Il Paese intero ha il diritto di conoscere come i propri amministratori impiegano le risorse pubbliche e con quali ricadute per il bene comune. un processo di responsabilizzazione sul fronte delle entrate: è stato giustamente osservato che non ci possono più essere centri di spesa totalmente deresponsabilizzati sul fronte delle entrate. poi affrontate seriamente le disuguaglianze territoriali in termini di sviluppo, di opportunità e di servizi che ancora dividono il Nord e il Sud del Paese. Un Mezzogiorno che deve accettare la sfida della responsabilità, della trasparenza, dell'autosviluppo, che intende scrollarsi di dosso sia la sindrome del risarcimento che quella del colonialismo, che si permette anche di ricordare al Paese che, se non recupera la sua unità sostanziale, rischia di essere nel suo insieme declassato dal novero dei quattro grandi Paesi europei: un destino che nessuno di noi, del Nord o del Sud, si deve augurare. È in questa direzione che dobbiamo accompagnare e completare le riforme strutturali che l'attuale Governo ha avviato: dal mercato del lavoro al nuovo *welfare* delle opportunità, dal federalismo fiscale ad un nuovo assetto della giustizia, dalla semplificazione degli apparati e dei procedimenti alla libertà di impresa, dalla scuola alla ricerca e all'innovazione come presupposto per accrescere il peso dell'Italia nell'Europa e nel mondo. colleghi, relatore, signora rappresentante del Governo, dobbiamo tutti insieme essere consapevoli che l'Italia ce la può fare attingendo alle sue virtù e alla sua genialità. Noi siamo chiamati ad offrire un contributo per dare più forza alle risorse vitali del nostro Paese, liberandolo da sprechi, inefficienze ed ingiustizie che si risolvono in una terribile ipoteca sulla qualità della vita odierna e sul futuro delle nuove generazioni. *(Applausi

capace di sviluppo e di crescita. Invece si sta discutendo di una manovra depressiva e iniqua, persino punitiva nei confronti di settori che sono per vocazione promotori di sviluppo e che per questo dovrebbero essere valorizzati, ma invece vengono mortificati.

il terzo l'occupazione femminile. A proposito di scuola, vorrei parlare degli insegnanti maltrattati e delusi, l'unica categoria che perde tre anni di attività lavorativa: vengono loro sottratti, e ciò si va ad aggiungere alla contrazione insostenibile del reclutamento, alla riduzione del numero degli insegnanti di sostegno, al fatto che quest'anno saranno alcune migliaia i bambini in lista di attesa, persino per la scuola dell'infanzia, che dovrebbe invece essere generalizzata, come è scritto in tutte le riforme approvate negli ultimi anni, fino ad una copertura vicina al 100 per cento della popolazione infantile. Quanto all'università, non ci sono segnali di ripristino delle risorse del Fondo ordinario, senza le quali - lo sanno tutti - il nostro sistema universitario sarà in ginocchio. Anzi, la manovra prevede ulteriori tagli, e avremo così scuola e università nelle condizioni dei Paesi più arretrati. Importanti enti di ricerca sono stati soppressi senza ragioni vere, con ricercatori umiliati: «potranno andare a fare altro», ci ha detto il Governo. poi le istituzioni culturali che vedono la voce relativa di bilancio ridotta del 50 per cento già da quest'anno, e dunque a progetti già avviati; per molti importantissimi istituti e fondazioni significa la chiusura. Tutto questo per risparmiare poche briciole,

Le fondazioni liriche si trovano in gravi difficoltà per gli effetti della conversione di un precedente decreto-legge. Insomma, signori del Governo e della maggioranza, state creando un deserto triste e cupo invece di considerare la cultura come una delle molle dello sviluppo del nostro Paese.

Ci sarebbe bisogno di politiche attive di sostegno all'occupazione e alla cura. Qual è, invece, la risposta del Governo per completare l'opera? Fare una cosa mai fatta per nessuno: aumentare in un solo colpo di quattro anni l'età pensionabile delle dipendenti pubbliche. Ma non è tanto questo il problema: è che ciò viene fatto senza dare loro adeguati riconoscimenti per la maternità e per la cura, senza adeguate e certe compensazioni in termini di servizi, di vantaggi fiscali, di accrediti figurativi per il periodo di maternità, come noi avevamo proposto. La sentenza della Corte europea è solo un pretesto per accelerare e prendere scorciatoie: questo è stato. Di fronte alle nostre proposte concrete avete girato la testa dall'altra parte; avete preferito un generico Fondo strategico in cui far confluire i risparmi senza certezze sulla loro reale destinazione. Magari si tratterà di briciole: lo vedremo.

*(IdV)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei anzitutto iniziare queste mie brevi considerazioni sul provvedimento in esame dalla vicenda che ha riguardato l'articolo 10 perché, al di là del merito, la ritengo la migliore rappresentazione del modo in cui Governo e maggioranza hanno affrontato tutta la manovra economica: una serie infinita di annunci, controannunci, smentite, rettifiche, in un balletto dal quale è emersa ancora una volta la totale mancanza di rispetto per l'istituzione parlamentare e per i cittadini. Tutto inizia con il Governo che presenta al Parlamento una norma che prevede un intervento di innalzamento addirittura di 11 punti (dal 74 per cento all'85 per cento) della soglia per l'invalidità civile. Tutto ciò al fine di raggranellare la ben misera cifra di 80 milioni di euro circa. Il 16 giugno, però, il senatore Gasparri annuncia a tutte le agenzie (leggo testualmente): «Voglio rassicurare in primo luogo le associazioni di categoria e tutti quanti pongono ancora oggi la questione della norma sulla soglia di invalidità. Non ci sarà alcun innalzamento della soglia dal 74 all'85 per cento per ottenere il diritto all'assegno di invalidità. Il Governo si è subito mostrato sensibile su questo punto e lo stesso ministro Tremonti ha dato il suo via libera perché questo punto della manovra correttiva sia cancellato». Peccato però che, invece di cancellare la norma, il 29 giugno sia stato presentato, a firma del senatore Azzollini, l'emendamento 12.1000 nel quale non solo continua pervicacemente a persistere l'innalzamento della percentuale di invalidità necessaria

limitando le future concessioni solo a chi è immobilizzato o non riesce a svolgere tutte le funzioni fisiologiche. Tale emendamento ovviamente scatena la protesta delle associazioni dei disabili, le quali giudicano subito la norma «largamente deludente e preoccupante (...), oltre che irridente a qualsiasi interlocuzione avvenuta e impegni assunti». Solo a questo punto il relatore annuncia un ulteriore emendamento soppressivo della norma sui criteri per l'invalidità civile. però, il livello di credibilità della maggioranza è ovviamente azzerato e perciò i disabili confermano la protesta che, infatti, si protrae fino all'annuncio della effettiva approvazione dell'emendamento soppressivo. Come ha scritto un autorevole osservatore: chi compenserà l'ansia e l'incertezza che migliaia di invalidi hanno provato in questi giorni? Chi è responsabile di tanta irriverente indifferenza nei confronti dei più deboli, camuffata da un indisponente atteggiamento da fustigatore di false invalidità? Ma il pasticcio delle pensioni di invalidità è solo uno dei tanti esempi del pressappochismo con il quale si è proceduto e si procede persino in materie così delicate come quelle sociali. Prendiamo, ad esempio, l'articolo 7, in cui si prevede la soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici. Tra questi, voglio soffermarmi su due casi in particolare: l'ISAE e l'ISPESL. Si tratta di due istituti diversi per funzioni: il primo si occupa di consulenza tecnico-scientifica in campo economico e della valutazione delle politiche economiche pubbliche; il secondo è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro. Ciò che li accomuna, tuttavia, è la riconosciuta competenza nei rispettivi campi e il prestigio - riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale delle personalità che all'interno di essi operano, esperti e validi ricercatori che sono membri attivi della comunità scientifica internazionale e che contribuiscono ad importanti progetti di ricerca. Nel complesso, secondo il Governo, i risparmi totali derivanti dal riassetto degli enti di previdenza sarebbero pari a circa 4,5 milioni di euro da riferire agli anni 2011 e successivi. Siamo certi che il risparmio di poche centinaia di migliaia di euro valga la perdita di un tale patrimonio di conoscenze e professionalità? In un Paese che già investe pochissimo nella ricerca e nella sicurezza sul lavoro sarebbero questi i grandi risparmi tanto pubblicizzati? E ancora, sempre a proposito di sicurezza sul lavoro, qualcuno è sinceramente in grado di spiegare quale sia l'utilità (e ancor di più la necessità) di una norma come quella contenuta nel comma 12 dell'articolo 8? Si prevede l'ennesima proroga dell'applicazione di una disposizione del decreto legislativo n. 81 del 2008, un testo che, peraltro, la maggioranza ha già provveduto a depotenziare ampiamente. La proroga dell'attuazione della normativa sullo stress da lavoro ed ancor più l'estensione della stessa al settore privato determinano un ulteriore segnale negativo per il Paese, mentre resta la domanda iniziale: quale sarebbe il vantaggioso effetto finanziario derivante da questa proroga? L'articolo 9 è un ulteriore e clamoroso esempio della fretta e dell'approssimazione con cui si è agito nella predisposizione di questo decreto. Una falcidia indiscriminata che colpisce in maniera orizzontale tutte le categorie del pubblico impiego, anche quelle già penalizzate da precedenti provvedimenti, peraltro - com'è stato maliziosamente notato - con una particolare attenzione, guarda caso, ad una delle categorie meno amate (soprattutto in questi giorni) dal Presidente del Consiglio. Se poi si leggono talune di queste disposizioni nel quadro complessivo della manovra si rilevano effetti paradossali. Mentre, ad esempio, si proclamano la guerra all'evasione fiscale e la caccia ai falsi invalidi, stabilendo a tal fine un programma straordinario di 100.000 verifiche per l'anno 2010 di 250.000 verifiche per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si inaspriscono ulteriormente le norme sul *turnover* nelle pubbliche amministrazioni. E tutto ciò in una situazione in cui l'INPS e l'INAIL non stanno neppure provvedendo ad assumere i vincitori di concorsi banditi ormai quasi 3 anni fa. Per quanto riguarda l'articolo 12, anche qui si possono riprendere le medesime considerazioni fatte all'inizio riguardo la vicenda delle invalidità. Anche su questo punto, infatti, l'*iter* è stato tutt'altro che lineare, con ripetuti e talvolta pasticciati interventi del Governo. Se anche fosse accettabile il fatto che un aumento dell'età pensionabile sia necessario, come sostenuto da più parti e in più occasioni e come espressamente richiestoci dall'Europa, ci si deve però chiedere perché si debba operare in regime di emergenza con provvedimenti *ad hoc*, che normalmente finiscono per essere iniqui perché vanno a toccare solo i pensionati di alcuni blocchi. La conseguenza è anche qui duplice: da un lato, sul piano politico, vi è il discredito di tutta l'istituzione parlamentare; dall'altro, sul piano pratico, come sempre l'effetto annuncio tende a vanificare buona parte dei risparmi, come già avvenuto nel 1992 e nel 1995. Nei periodi precedenti le riforme si verifica infatti solitamente un'impennata nel numero delle uscite per pensionamento. In questo caso, l'effetto congiunto del ritardo delle finestre e della rateizzazione del trattamento di fine rapporto (di cui al comma 7) saranno un forte incentivo a scappare appena possibile. II comma 10 del medesimo articolo 12 stabilisce che, dal 1° gennaio 2011, a tutte le buonuscite dei dipendenti pubblici si applicherà il meccanismo di calcolo che regola il trattamento di fine rapporto nelle aziende private. Tale novità non è retroattiva ed opera *pro rata* sulle *tranches* di liquidazione *post* 2011, ma, una volta a regime, l'equiparazione con i privati potrebbe essere solo teorica e nascondere qualche insidia in più per chi lavora nella pubblica amministrazione. Le nuove norme riguarderanno quasi esclusivamente i dipendenti pubblici, che finora contavano di concludere la loro carriera con una buonuscita calcolata in rapporto all'ultima retribuzione annua. L'unità di misura per l'assegno di questi dipendenti è infatti l'80 per cento delle voci fisse lorde dell'ultimo anno, divise per 12. Tuttavia, ora l'ancoraggio della liquidazione alla retribuzione finale viene abbandonato e a ciò va aggiunto l'elemento, ben più pesante, del fatto che il TFR dei lavoratori privati abbraccia come base di calcolo quasi tutta la busta paga, mentre negli uffici pubblici contano per il calcolo della buonuscita solo le voci fisse (le voci variabili sono ininfluenti). Di fatto, dunque, l'equiparazione delle regole per le liquidazioni tra settore privato e settore pubblico rischia di essere solo nominale, o addirittura di creare forti disparità. A ciò si aggiunga che, alla luce delle recenti riforme del pubblico impiego, è proprio il peso delle voci stipendiali variabili ad essere destinato ad assumere sempre maggior rilievo. Come già detto, il cambio di regole potrebbe spingere ad anticipare l'uscita di molti dipendenti pubblici che hanno i requisiti per farlo. Ancora una volta, insomma, stiamo navigando a vista. E intanto tutti gli istituti nazionali ed internazionali ci segnalano una situazione economica stagnante e soprattutto una disoccupazione a livelli record,

chi parla di crisi viene bollato di pessimismo e di disfattismo, seguono rapidamente periodi in cui esplodono le emergenze e dunque si deve agire in fretta. E la fretta, mai come in questo caso, è cattiva consigliera.

soltanto alcuni *flash*; è infatti impossibile - e mi sembra anche inutile - discutere in quest'Aula assolutamente vuota e con l'annunzio di una fiducia che, secondo un sistema ormai scandito, si ripete continuamente. La manovra sottoposta all'Aula del Senato, senza sostanziali variazioni dello schema iniziale, non consente al nostro sistema produttivo di affrontare le difficoltà indotte dalla crisi economica e finanziaria in corso. Se questo è il contesto, non è possibile ignorare che la tutela giurisdizionale, nella sua efficienza, rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese. La competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali si favoriscono difatti anche con procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali e con il contrasto ad attività scorrette ed illegali, che alterano le regole di mercato e della concorrenza. Ebbene, il sistema giudiziario italiano soffre di gravi carenze strutturali, che il Governo non intende affrontare con una effettiva organica riforma, pur sollecitata da tutti gli operatori della giustizia, ma che anzi dimostra di voler aggravare con la esiguità degli stanziamenti economici assegnati alla giustizia. Ne è prova l'ultima manovra finanziaria, che ha ulteriormente ridotto le risorse stanziate rispetto all'esercizio precedente, ove già rappresentavano soltanto l'1,4 per cento del bilancio dello Stato. oggi il Governo aggiunge al taglio di oltre 327 milioni di euro operato nel corso della precedente finanziaria, il taglio di altri 140 milioni di euro nel triennio alla missione 6 (Giustizia). Una riduzione significativa e suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello standard qualitativo dell'amministrazione della giustizia, se solo si considera che a tale missione sono riconducibili quattro programmi cruciali per la funzionalità della giustizia e quindi anche per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini - come quelli della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell'amministrazione penitenziaria, nonché dell'edilizia penitenziaria e minorile. Una riduzione che vuole ignorare che nell'ultimo anno si è registrato un incremento significativo delle morti in carcere e dei suicidi di detenuti, di cui sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e la carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale, conseguenza di un incremento preoccupante del sovraffollamento negli istituti penitenziari, fatto per cui l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'articolo 3 della Quindi, la manovra appare assolutamente inefficace e il Governo, a fronte della continua introduzione di nuove norme incriminatrici, spesso riferite a condotte prive di offensività giuridica, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, con il rischio (che probabilmente a questo punto dobbiamo ritenere calcolato) di minare la certezza del diritto e la credibilità della funzione giurisdizionale, senza curarsi dei gravi pregiudizi per la sicurezza e la tutela dei diritti dei cittadini. Si ostacolano infatti la piena attuazione di politiche per la sicurezza e il contrasto alla criminalità, impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati e l'identificazione dei colpevoli, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto asserito da esponenti di Governo e maggioranza non solo in sede parlamentare e in contesti istituzionali, ma anche nella comunicazione costantemente reiterata attraverso gli organi di stampa. Se questo è l'intento, si comprende perché Governo e maggioranza non prestino attenzione né ai suggerimenti dell'opposizione né a quelli degli operatori della giustizia. Cade inascoltata, ad esempio, la protesta dell'avvocatura italiana, che sottolinea come la crisi economica non può essere il pretesto per tagliare ulteriormente le risorse alla giustizia. Inutile ovviamente anche la protesta del personale amministrativo. Parole inutili in un Paese in cui il *Premier* ed esponenti di Governo cercano costantemente di convincere l'opinione pubblica a considerare giustizia e pubblica amministrazione non una risorsa, ma un costo addirittura uno spreco. Tutto ciò risponde ad una logica: è più facile, in questo modo, incidere negativamente su giurisdizione e pubblico impiego, evitando di colpire gli evasori fiscali (già beneficiati da numerosi condoni e scudi fiscali), i patrimoni illeciti, le grandi rendite e le ricchezze del settore privato; paralizzando l'intero sistema giudiziario, screditando e mortificando il personale amministrativo; svilendo la dignità della funzione giudiziaria e cercando, per quanto possibile, di minarne l'indipendenza, l'autonomia, il rilievo costituzionale, l'autorevolezza. Signora Presidente, io invece leggerò il mio intervento, perché voglio che rimanga agli atti della discussione che avviene dopo le note e iperdiscusse vicende di cui la Grecia ha rappresentato l'epifenomeno. Il Parlamento si appresta ad approvare, attraverso l'ennesima fiducia per esigenze tutte interne alla maggioranza, la manovra che dovrebbe essere in linea con quanto anche il Governo italiano ha discusso ed approvato in sede europea e - vorrei farlo presente al presidente Azzollini - non solo nel vertice europeo del maggio scorso. Dopo tale vertice c'è stata, infatti, una riunione del Consiglio europeo per definire la nuova strategia di superamento della crisi. Ci saremmo aspettati di discutere di una manovra che avesse almeno qualche punto di corrispondenza con quanto si sta facendo in tutta l'Unione europea. Così non è, perché i tagli che si propongono, oltre ad essere iniqui, non assicurano la coerenza con gli obiettivi strategici europei, che certamente contemplano il contenimento della spesa pubblica, ma guardano anche a interventi di sostegno della crescita. crescita. La nuova strategia messa a punto dal Consiglio europeo, in data 17 giugno, è infatti una strategia per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Ricordo a tutti noi che il documento approvato in sede di Unione europea recita: «La strategia aiuterà l'Europa a riprendersi dalia crisi e ad uscirne rafforzata, a livello sia interno che internazionale, incentivando la competitività, la produttività, il potenziale di crescita, la coesione sociale e la convergenza economica. La nuova strategia risponde alla sfida di riorientare le politiche per passare da misure di gestione della crisi all'introduzione di riforme a medio-lungo termine volte a promuovere la crescita e l'occupazione e ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, tra l'altro anche attraverso la riforma dei sistemi pensionistici». «il miglioramento del potenziale di crescita dovrebbe essere considerato fondamentale per agevolare il risanamento dei conti pubblici a lungo termine». Nulla, Presidente, nulla di quanto contenuto nella manovra va in questa direzione: non incentivi a produttività e competitività, zero strategia per la crescita e quanto alla coesione sociale, ricordando che l'Italia è il terzo Paese ad usufruire dei fondi europei per la coesione, c'è da chiedersi in che modo il Governo intenda procedere con il cofinanziamento necessario per l'attivazione dei medesimi, cosa che si è chiesto anche il commissario europeo alle politiche di coesione nel corso dell'audizione che ha recentemente tenuto nel Parlamento italiano. Vede, Presidente - parlo solo con lei - il problema che noi poniamo non è sull'entità dei tagli certamente in linea con quanto richiesto da Bruxelles; quello che non quadra - e qui Bruxelles non entra nel merito perché sono scelte nazionali - sono gli obiettivi dei tagli: tutti a carico di chi già paga gravemente la crisi. Ora, l'Italia è caratterizzata per un livello dei salari tra i più bassi di Europa e per una forte accentuazione delle diseguaglianze sociali. Ed era già così prima della crisi i signori della maggioranza, in due anni di Governo, non hanno fatto niente per ridurne le conseguenze negative soprattutto per i più bisognosi. Non è una forzatura quindi sostenere che ormai nel nostro Paese la classe media è ridotta quantitativamente ai lumicino. In tale situazione lo strumento fiscale deve tornare a svolgere un ruolo attivo nel senso dell'equità e della progressività. D'altronde, è largamente diffusa nella pubblica opinione la consapevolezza di una non più sostenibile divaricazione delle condizioni economiche e sociali. Tra le altre cose, i dati OCSE 2008 ci ricordano che la percentuale di gettito proveniente da imposte patrimoniali è pari a 4,3 in Italia, a 10,2 in Canada, a 7,8 in Francia, a 15,1 in Giappone, a 11,7 negli USA e nel Regno Unito. Aggiungo, se fosse necessario ancora sottolineare come si allarghi la forbice che ci divide dal resto dell'Europa, che il Consiglio europeo ha fissato cinque obiettivi principali, oggetto di un nostro ordine del giorno, che riguardano incentivi per l'occupazione femminile, interventi a sostegno della ricerca e dello sviluppo, misure a favore della *green economy*, sostegno all'istruzione e alla formazione, inclusione sociale e lotta alla povertà. Ed è bene ricordare, a chi dai banchi della maggioranza chiede una *governance* europea più forte, che nelle manovre attualmente in approvazione nei diversi Paesi europei si ragiona sia su nuovi strumenti fiscali sia sul carattere progressivo dell'imposta sul reddito. Solo per fare qualche richiamo: dalla Germania che introduce una tassa ecologica sui voli aerei (1 miliardo il gettito previsto) e un'imposta sull'attività bancaria (2 miliardi dal 2012), alla Spagna dove diverse Regioni prevedono l'innalzamento dell'aliquota marginale dell'imposta sul reddito cento sopra ai 120.000 euro e al 47 per cento sopra a 175.000 euro di reddito annuo. A chi sostiene la politica dei due tempi prima i conti pubblici e poi la crescita - perché questo non sarebbe il momento politicamente opportuno per affrontare le tematiche, indubbiamente delicate, che la crescita pone, non si può non rivolgere la classica domanda: se non ora, quando? Vedete, cari colleghi della maggioranza, il punto è che queste tematiche devono essere affrontate nell'interesse generale del Paese e per il futuro dell'Europa. Sulla maggioranza pesa la responsabilità maggiore del rispetto delle regole comuni, come nel caso delle quote latte, e per cortesia non utilizzate facili e dannose scappatoie, come quella di continuare a dire all'opinione pubblica «facciamo la manovra perché ce lo impone l'Europa», perché in questo modo fate diventare l'Europa sempre più impopolare tra i cittadini. Il problema non è l'Europa, ma la politica di questa maggioranza, la politica economica e sociale di questo Governo, la sua concezione della gestione della cosa pubblica, la sua idea di una Europa intergovernativa a discapito di quella comunitaria. Queste sono ragioni molto concrete che sollevano molti fronti di protesta perché si tratta di diritti essenziali dei cittadini sui quali c'è bisogno di condivisione e non certo di imposizioni. Per questo respingiamo le accuse di irresponsabilità di fronte ai problemi difficili dell'Italia e dell'Europa e ribadiamo che quello che ci interessa è il merito delle questioni economiche e sociali, di cui vogliamo discutere con lungimiranza ed equilibrio. Nient'altro. Per noi, oggi più che mai, è inevitabile che sia così, perché ne hanno bisogno la nostra democrazia, la rete dei poteri regionali e locali, la sfera della rappresentanza, il sistema economico e delle garanzie. Ed è perfino superfluo ricordare che ne ha bisogno l'appartenenza e il ruolo dell'Italia nell'Unione europea e nel mondo.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, possiamo dire in tutta tranquillità che il provvedimento oggi al nostro esame ha un titolo inequivoco e molto chiaro: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». Questo provvedimento contiene quindi misure per la stabilizzazione finanziaria - ossia contiene impegni assunti in sede comunitaria sulla stabilità finanziaria del nostro Paese e misure per la competitività economica. Ovviamente, le misure per la stabilizzazione finanziaria sono una precondizione per l'attuazione delle misure di sostegno e di rilancio della nostra economia. Viviamo in un momento cruciale per l'economia dell'area euro e del nostro Paese e sappiamo tutti che ci troviamo nella peggiore recessione degli ultimi 80 anni. però qualcosa di peggiore della recessione, ed è la bancarotta dello Stato. Senza questa manovra, le possibilità di insolvenza del nostro Paese aumenterebbero in maniera esponenziale. Quelli contenuti in questa manovra sono indubbiamente sacrifici severi, che si impongono se vogliamo evitare il rischio Grecia o il *default* argentino. Le difficoltà dell'Argentina, e poi, soprattutto, della Grecia non costituiscono, come abbiamo appurato, un fenomeno circoscritto. Ecco perché si è deciso, concordemente agli altri Paesi dell'area euro, di ripristinare il pieno controllo sui saldi di bilancio pubblico. I Paesi dell'area euro stanno tutti adottando manovre pesanti, lo si è ribadito anche oggi in quest'Aula. La Francia sta discutendo una manovra da 100 miliardi di euro, la Germania da 45 miliardi di euro, e noi stiamo adottando una manovra correttiva da 25 miliardi di euro, che intende ridurre i saldi di finanza pubblica nei prossimi due anni. La dimensione è quella minima necessaria per riportare sotto controllo le finanze pubbliche. Questa è la ragione per la quale la manovra di questo Governo è stata accolta con favore dai Ministri delle finanze dell'area euro. La linea del rigore oggi non ha alternative e nel medio-lungo periodo renderà più solida e duratura la crescita economica. tagli alla spesa pubblica e il contrasto all'evasione fiscale e contributiva sono le sue macroaree di intervento. La manovra è stata perfezionata grazie al sapiente lavoro della Commissione bilancio

Sul versante del contenimento della spesa pubblica, la manovra spiega indubbiamente i suoi effetti più forti. Ridurre la spesa pubblica è un dovere morale se vogliamo liberare risorse destinate alla crescita e abbassare la pressione fiscale in futuro. La manovra si concentra per circa due terzi del totale sulla riduzione delle spese e i tagli sono concentrati sulla spesa corrente. Certo, la manovra incide anche sul comparto delle autonomie locali, ma sono stati introdotti criteri di differenziazione di virtuosità nel taglio delle risorse al comparto delle autonomie. Per le autonomie locali c'è poi un impegno assunto dal Governo che ci tranquillizza, anche come amministratori locali: entro il 31 luglio dovrà essere presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo sull'autonomia fiscale degli enti territoriali e entro il prossimo anno verranno rivisti i parametri del Patto di stabilità. Le esperienze di gestione del Patto a livello regionale potrebbero costituire una preziosa base di riferimento. Una gestione del Patto di stabilità su scala territoriale consentirebbe di ridurre la rigidità del sistema e di ottimizzare la ripartizione delle quote di indebitamento tra amministrazioni locali. Abbiamo poi particolarmente apprezzato l'eliminazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali: si tratta di un organismo inutile e ormai votato solo alla sterile difesa corporativa di una categoria che deve essere ripensata radicalmente. Speriamo che questa eliminazione possa resistere fino a domani mattina, quando ci sarà la presentazione del maxiemendamento. La strategia di contrasto dell'evasione proposta da questa manovra va nella giusta direzione, ossia verso l'anticipo di un fisco federale, rilanciando il ruolo dei Comuni nell'attività di accertamento fiscale, prevedendone una specifica collaborazione con l'Agenzia delle entrate e disegnandone un ruolo propulsivo nei confronti dell'Agenzia del territorio, ai fini dell'aggiornamento del catasto e dell'individuazione degli immobili non dichiarati al fisco. Grazie ai Comuni, finalmente la lotta all'evasione potrà essere selettiva e non colpirà nel mucchio, come oggi, purtroppo, accade spesso. Il funzionamento di questo nuovo meccanismo sarà legato alla sensibilità politica dei Comuni, alla preparazione dei funzionari comunali incaricati di questa delicata attività di accertamento, ma anche e soprattutto alla collaborazione delle Agenzie delle entrate e del territorio. Vogliamo ribadire che, superata questa manovra correttiva, la strada maestra per noi è e rimane quella del federalismo fiscale e istituzionale. Qualcuno sostiene che questa manovra metta un seria ipoteca sul processo di attuazione del federalismo fiscale. La realtà è che questa manovra correttiva, frutto di un vecchio e vigente regime di finanza derivata fatto di trasferimenti dello Stato e di conseguente irresponsabilità dei centri di spesa, ci fa comprendere quanto sia necessario attuare il federalismo fiscale e dare autonomia e responsabilità agli enti locali. In questo quadro parlare di Ministeri in Padania non significa parlare di un sogno irrealizzabile, ma della doverosa distribuzione territoriale delle articolazioni di Governo. Accanto ad una distribuzione federalistica della sovranità fiscale deve verificarsi una distribuzione federalistica della sovranità istituzionale. Pensare Milano (capitale economica di questo Paese), oppure Torino (capitale morale di questo Paese), oppure Venezia (capitale culturale di questo Paese) come sedi di Ministeri o di Autorità importanti non significa lanciare una provocazione estiva, ma seguire la linea democratica che in altri Paesi è già stata ampiamente perseguita, se vi è l'effettiva volontà di trasformare l'assetto istituzionale del nostro Paese in uno Stato federale. L'Europa vive oggi una fase delicata e non solo per le finanze pubbliche e per i destini della moneta comune; soffia un vento di riforme costituzionali in Belgio, in Spagna (dove il 48 per cento dei catalani si dichiara a favore della secessione) ed in Scozia. Proprio in Scozia, dopo la *devolution* voluta da Blair nel 1999, si discute democraticamente e pacificamente del metodo per raggiungere l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito, la politica scozzese si divide tra i gradualisti e i fondamentalisti, che hanno come elemento distintivo solo il modo per raggiungere il comune obiettivo dell'indipendenza. Gli scozzesi lamentano di dover sopportare un carico fiscale eccessivo rispetto al resto della comunità in cui si trovano inseriti e quindi chiedono di secedere; l'analogia con la circostanza in cui si trovano le Regioni del Nord è a noi tutti evidente. Noi non siamo per la logica del tanto peggio tanto meglio, ed è per questo che votiamo in maniera convinta questa manovra correttiva. Vorremmo condurre questo Paese fuori dall'emergenza finanziaria e poi concordare democraticamente i passaggi necessari e l'obiettivo finale del nostro movimento, che è e rimane la libertà e l'indipendenza della Padania, un federalismo come assetto stabile per riconoscere, tutelare e gestire le diversità. Il diritto alla nostra diversità non può più essere negato senza innescare il ricorso al rimedio ultimo, o alla risorsa estrema, come diceva Gianfranco Miglio, del diritto alla secessione.*(Applausi

Signora Presidente, a differenza di quanto si è affannato a dire il ministro Fazio, il taglio sulla spesa sanitaria c'è e farà sentire i suoi effetti nefasti quanto prima. Altri Paesi europei hanno fatto delle manovre anche più pesanti della nostra, ma hanno inserito degli elementi di rilancio dell'economia e, fra questi, quelli per la sanità, la ricerca e la scuola. Ciò, in piena sintonia con l'Europa che, nella strategia per la salute 2008-2013, ha puntato sulla promozione della salute come fattore decisivo non solo per il benessere degli individui e della società ma anche come prerequisito per la produttività e la prosperità economica. Da noi, invece, alle Regioni viene richiesto un taglio così drastico di risorse che non potrà non incidere sui bilanci della sanità, che rappresentano oltre l'80 per cento del totale delle risorse dei loro bilanci. Da mesi ci sentiamo dire che il federalismo e i costi standard sono la chiave di volta per l'uscita dalla crisi del sistema Paese, e poi la prima cosa che la maggioranza fa è stracciare unilateralmente il Patto per la salute sottoscritto, dopo mesi di scontri durissimi tra le Regioni e lo Stato, tra le Regioni e lo Stato, solo nel dicembre scorso. Il Patto per la salute è lo strumento pattizio che ha consentito in questi anni di dare un ruolo alle Regioni nella programmazione e nel controllo della spesa sanitaria. La sanità è l'unica vera materia dove si è pienamente esercitato il federalismo regionale. Le Regioni hanno più volte denunciato in questi giorni i punti in cui la manovra ha violato il Patto per la salute; ne citerò solo due. i 550 milioni di euro che erano stati previsti essenzialmente per l'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (perché noi siamo fermi a quelli del 2001), che naturalmente sono stati tagliati, per cui rimangono solo 300 dei 550 milioni di euro promessi, e anche questi ipotetici, perché subordinati ad economie in campo farmaceutico. Questo dopo che, per anni, il Ministro e i membri della maggioranza hanno promesso agli ammalati di malattie rare, di SLA, di malattie croniche che i nuovi LEA erano sulla dirittura d'arrivo, mentre con questa manovra sui LEA cade una pietra tombale.

che erano stati tagliati dopo quelli proposti dal Governo Prodi, oggi siamo di nuovo daccapo. Siamo convinti della necessità della manovra, ma ne contestiamo i contenuti, in particolare, nel settore della salute. In primo luogo, perché il nostro sistema sanitario è tra quelli europei che costa meno (il 6,9 inoltre, perché i tagli orizzontali che si sono perseguiti non riducono strutturalmente la spesa e non aiutano a ricodificare i servizi. L'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali in un recente convegno tenuto presso la biblioteca del Senato ha richiamato la nostra attenzione su alcuni indicatori di *performance* dei sistemi sanitari regionali, che riguardano: il tasso dei ricoveri, il tasso di ospedalizzazione e la percentuale di anziani assistiti a domicilio. Ebbene, nelle realtà non virtuose addirittura il 40 per cento dei pazienti viene nuovamente ricoverato entro 30 giorni dalle dimissioni. In queste stesse realtà il tasso di ospedalizzazione è maggiore del 18 per cento e circa il 50 per cento degli anziani non può godere dell'assistenza domiciliare andando ad incrementare il numero dei ricoveri in proprio. Sono queste le questioni che andavano aggredite, e non operare i tagli orizzontali

Da ciò emerge che il raggiungimento di parametri virtuosi può incidere non solo sul livello della spesa, ma anche sulla qualità delle cura e sugli obiettivi salute del nostro Paese. salute del nostro Paese. Questo ci dice che investire in modo selettivo in salute, premiando le azioni virtuose, non solo riduce i costi ma aumenta il PIL ed i diritti dei cittadini, mentre una manovra siffatta servirà solo ad inasprire il rapporto con le Regioni, a danneggiare il diritto alla salute, a non modificare in modo strutturale la spesa e, inoltre, a colpire professionalità e competenze.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, la manovra economica alla nostra attenzione ha suscitato vaste proteste nel Paese. Seppur necessaria per contrastare la crisi economica attraverso il riordino dei conti pubblici, si abbatte però in modo indiscriminato sui ceti popolari e, in particolare, sulle categorie più povere ed indifese. Si chiede ai cittadini di tirare la cinghia, di risparmiare anche sul necessario, ma non si creano le condizioni per uscire in positivo dalla recessione

il nostro è l'unico Paese che affronta questa emergenza senza un Ministro dello sviluppo economico, senza quindi una guida dell'economia reale. Questa inettitudine di carattere strategico è particolarmente evidente nell'assenza di una seria politica di innovazione del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione. In tutti i Paesi sviluppati i Governi hanno messo in campo politiche volte ad innovare il sistema delle comunicazioni attraverso la diffusione della banda larga. Tutti lo hanno programmato, nella convinzione generale che questa innovazione di sistema può creare nuovo lavoro nell'immediato e, soprattutto, può contribuire grandemente alla risalita del PIL. Il professor Mario Monti, nel suo recente *report* al presidente Barroso sul rilancio del mercato unico europeo, afferma che l'Unione europea potrebbe aumentare il suo PIL del 4 promuovendo il mercato unico digitale entro il 2020. Questo incremento corrisponde a 400 miliardi di euro"! Ripeto, 400 miliardi. Per Per fare ciò occorre un grande piano per l'economia digitale, a partire dall'implementazione dell'infrastruttura di rete, con l'obiettivo di portare entro il 2013 la banda larga a tutti gli italiani e, entro il 2015-2020, alla costruzione di una rete di prossima generazione, la cosiddetta banda ultralarga. Sono questi gli obiettivi dell'Agenda digitale europea di recente avviata in sede comunitaria. Francia, Germania, Inghilterra sono su questa lunghezza d'onda. L'Italia è al palo. Il piano Caio si è trasformato in piano Romani; si è portato il tutto al CIPE e da lì non è più uscito nulla. Intanto, gli 800 milioni di euro di dote sono scomparsi nei mille rivoli della spesa corrente. Quel piano, pur modesto, poteva generare almeno 50.000 nuovi posti di lavoro e dare impulso al mercato per altri più corposi investimenti, con l'obiettivo di abbattere il *digital divide* e di realizzare la più importante innovazione del Paese in questo inizio di XXI secolo. La banda larga non è solo un potente stimolo alla crescita economica del sistema produttivo,

Signori del Governo, voi rinunciate a tutto ciò. A voi non importa nulla del futuro del Paese. Non solo avete colpevolmente bloccato i vostri stessi piani di investimenti sulla banda larga, ma rinunciate anche al "tesoretto" delle frequenze dello spettro radio che si liberano nel passaggio dalla vecchia televisione analogica a quella digitale terrestre. È il cosiddetto dividendo digitale. Parliamo di un bene pubblico di valore notevole che la Commissione europea, con la decisione del 6 maggio 2010, ha chiesto agli Stati membri di mettere a disposizione per i servizi di comunicazione mobile a banda larga. Colleghi, tutti gli Stati più attenti alle nuove tecnologie stanno provvedendo, mettendo a gara pubblica le frequenze. In Germania il Governo ha già incassato 4,5 miliardi di euro; in India 8,3 miliardi.

Con queste risorse si può realizzare il piano Romani e fare, quindi, investimenti per la crescita economica. E ne avanzano per evitare di fare *tabula rasa* degli enti culturali o di fare scempio dei diritti degli invalidi ad avere un sostegno adeguato da parte dello Stato.

Lo abbiamo ripresentato in Aula con caparbietà, e lo ripresenteremo anche alla Camera se non verrà compreso nel maxi emendamento del Governo. Non buttiamo al vento questa grande opportunità di innovazione e di crescita. Non regaliamo un bene pubblico prezioso. Non dissipiamo per il solito conflitto di interessi risorse rilevanti per il bilancio dello Stato. Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, assumo il contenuto di questo disegno di legge come un documento con finalità altamente pedagogica: educare noi stessi, educare gli italiani, educare l'apparato pubblico e privato alla sana e razionale amministrazione. È un'attività che, se l'avessimo intrapresa prima, probabilmente oggi non avremmo il peso che abbiamo e la necessità di adottare provvedimenti restrittivi del tipo di quelli al nostro esame. Dico ciò perché già negli anni Ottanta, all'alba della riforma della sanità, si diceva questo Paese non poteva più reggere il peso notevole dell'apparato pubblico, dello Stato sociale, che pure avevamo perseguito e conseguito ma che si appalesava tanto sclerotizzato da avere bisogno di ammodernamento e di efficientizzazione. In fondo, i titoli delle partizioni di questo provvedimento di riduzione del perimetro dei costi della pubblica amministrazione, quindi di un'opposizione alla dequalificazione della spesa con utilizzo di stanziamenti in conto capitale per finalità che sono di spese correnti. Non è da oggi ma da 15 anni che la Banca d'Italia va predicando la necessità di contrarre la spesa corrente e di spingere sulla spesa per investimenti. Conteniamo il costo di funzionamento dello Stato e degli enti locali, sopprimiamo gli enti inutili, razionalizziamo e risparmiamo sulla spesa della pubblica amministrazione e, perché no, anche della spesa sanitaria. Chiunque provi a passare tra gli ospedali italiani non può non rilevare che molti di essi, molti reparti, si rivelano essere realtà assimilabili ad un albergo più che a luoghi di cura. di cura. Questo provvedimento, che va in direzione di contenere la spesa, di finalizzarla e qualificarla, deve spingere tutti quanti, operatori e non, utenti ed applicati, dipendenti della pubblica amministrazione ed operatori privati, a prendere atto che le risorse che si assumono per la via della tassazione meritano certamente una migliore erogazione e una migliore finalizzazione.

ci può mettere nelle condizioni di affrontare un nuovo compito, e in quella fase di novità e di nuova applicazione, probabilmente si potranno produrre risultati che non siamo riusciti a produrre con l'Italia delle autonomie nell'ultima fase della sua applicazione.

che se non ci fosse questa malapianta probabilmente avremmo uno sviluppo economico corrispondente al doppio dell'incremento di PIL che si è verificato negli ultimi anni in Italia, in generale, e nel Mezzogiorno, in particolare. Fermo restando che dobbiamo essere consapevoli che di questi provvedimenti probabilmente ne dovremo adottare altri, perché il tunnel non ci consente ancora di vedere la luce, guardiamo con interesse ai fondi strutturali

guardare alla rivitalizzazione dei centri storici, che significa "edilizia". Va bene infatti la banda larga, della quale non ci dobbiamo scordare, ma la qualificazione del personale e dei lavoratori italiani vuole una risposta immediata,

della chiave di partenza potrebbe consentire di riprendere il percorso di questo Paese, più segnatamente, delle aree che abbisognano di sviluppo e di occupazione, anche nella logica di contenere lo sviluppo della criminalità che corre in misura più veloce rispetto ai pur grandi risultati che, grazie alle forze dell'ordine e alla magistratura, il Paese sta conseguendo. Si guardi allora immediatamente alle infrastrutture. Ognuno di noi faccia la propria parte per convincere gli italiani, e noi innanzitutto, che abbiamo bisogno di subire un lungo percorso di esame e di riconsiderazione della spesa pubblica, poiché le Befane non ci sono più, e ciò ci mette nelle condizioni di prendere atto che non è soltanto una condizione nostra, ma riguarda tutte le economie mature, tutti i Paesi d'Europa per quanto ci sono più vicini.

perché bisogna farne altri se si vuole essere leali con sé stessi e con il Paese, atteso che molto a lungo abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità e abbiamo utilizzato risorse in misura superiore a quelle che abbiamo prodotto. Non si trascuri tuttavia l'utilità della spesa dei fondi strutturali, che soli possono consentire di perseguire e conseguire il riequilibrio territoriale, che è il primo obiettivo

la qualità alberghiera dei nostri ospedali è ancora ben lungi dall'essere ottimale in tante Regioni italiane; peraltro, in questa manovra non se ne fa menzione.

politica e personale. Se fossimo in un momento di ordinarietà della situazione economica internazionale, con un'Europa forte e il nostro Paese in forte crescita potrei dire che questa manovra,

in un quadro europeo debole e di instabilità complessiva, accompagnare questa situazione semplicemente con tagli di costi e della spesa pubblica mi sembra veramente una scelta miope.

hanno abbandonato la frontiera del separatismo padano e probabilmente si sono accomodati al più confortevole ristorante del Senato, ma vorrei dir loro che agitando la bandiera del federalismo e della separazione non risolviamo in questo momento i problemi degli italiani. Probabilmente il federalismo fiscale ci serve per rendere efficiente un sistema ed una società: ma qual è il modello di società che vogliamo? Noi, come Partito Democratico, proponiamo un modello di società solidale, un nuovo modello di coesione sociale

insieme il Paese. La manovra rischia di colpire proprio la classe media, una classe media che tende ad assottigliarsi sempre di più. Ciò significa che da una parte aumentano i ricchi e dall'altra aumentano i poveri,

che precede l'imposizione del voto di fiducia per l'approvazione della manovra economica. Mi limiterò a segnalare alcuni aspetti assurdi di questa vostra manovra, con particolare riferimento al tema della sicurezza, a quello della giustizia e alla materia concernente la sicurezza sul lavoro. Ad onta di tutto quello che il Governo, *in primis* il ministro Maroni ed il ministro Alfano, continua a dichiarare agli organi di stampa e alle televisioni sulla priorità delle questioni attinenti alla sicurezza dei cittadini e al collegato problema del sistema giustizia, assiste per la terza volta ad una rinnovata mannaia che viene calata brutalmente, ma chiaramente, sulle necessità e le esigenze delle nostre forze di polizia e sulle correlate necessità della macchina della giustizia, già tanto ingolfata e ormai ai limiti del collasso. Le cifre sono evidenti nella loro negatività, e non si tratta di tagli e blocchi delle spese legati alla grave crisi economica interna ed internazionale perché già nel luglio di due anni fa voi, signori del Governo, avete approvato un Documento di programmazione economico-finanziaria che nei tre anni a venire prevedeva tagli di circa il 40 per cento, sia per il comparto sicurezza che per il sistema giustizia. E ciò lo avevate fatto ancor prima della crisi finanziaria mondiale, considerato che il fallimento della società americana Lehman Brothers risale alla metà di settembre di due anni fa. Ciò significa ancora che voi, sedicenti paladini della sicurezza dei cittadini e dell'ordine, avevate programmato fin dall'insediamento del vostro Governo tagli, tagli e ancora tagli ai danni di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e magistratura. Tagli e tagli che continuate a fare anche oggi, rigettando i nostri emendamenti, nonostante le pesanti contestazioni che ormai tutti gli operatori della sicurezza, quelli che lavorano sul campo ogni giorno, tutti i sindacati di polizia, di destra, di centro e di sinistra, vi rivolgono, senza distinzioni di colore politico, accomunati solo dalla consapevolezza che voi state distruggendo in Italia il sistema della sicurezza dei cittadini, state finendo di demolire ogni parvenza di sistema giudiziario. In compenso, quel che vi sta a cuore e vi ossessiona è soltanto di impedire che le indagini di polizia e magistratura possano giungere ad un processo che accerti i crimini della "cricca", che affermi le vostre responsabilità, oltre che politiche, anche penali. Così come vi tormenta una libera stampa che dia, per dovere costituzionale, informazioni e notizie corrette sul vostro amorale modo di intendere la politica: alla faccia dei tanti proclami leghisti e dei vostri Ministri dell'interno e della giustizia! Alla faccia della legalità costituzionale! Vi è un altro aspetto della vostra manovra economica che voglio considerare. È quello relativo alla soppressione dell'ISPESL, istituto avente competenze fondamentali in materia di sicurezza dei lavoratori. Ora voi, con la copertura di un intento riformista (peraltro falso riformismo liberista), in realtà continuate nella vostra politica di eliminare dall'ordinamento qualsiasi tipo di controllo di sicurezza industriale degli insediamenti produttivi e nei luoghi di lavoro. In pratica, con questa vostra sorta di criptoriforma, abrogativa della riforma sanitaria nella parte concernente la prevenzione e quindi la sicurezza sul lavoro, disponete l'accorpamento dell'ISPESL all'INAIL (operazione già di per sé illogica e contraddittoria), ma vi dimenticate, non casualmente, di garantire le funzioni dell'ISPESL di verifica della sicurezza degli impianti e degli apparecchi sui luoghi di lavoro, oltre che le funzioni concernenti la consulenza e i pareri allo Stato in materie importantissime, quali quelle sugli standard dei prodotti industriali, sulla produzione, impiego e commercio di sostanze chimiche e di energie capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico, sui controlli sanitari in materia di energia nucleare e sostanze radioattive, sulla disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Procedendo a questa sorta di controriforma, non vi peritate nemmeno di considerare che la soppressione dell'ISPESL

Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi non è certo facile per i rappresentanti della Valle d'Aosta, cioè di una Regione a Statuto speciale con più di 60 anni di storia di federalismo - e non solo di quello fiscale - che vuole comunque collaborare per far crescere tutto il Paese, definire positivo il testo di una manovra che prevede un ingente prelievo economico alle Regioni. È difficile definire positiva una misura che ha tra i suoi obiettivi principali, almeno nel testo iniziale, quello di ridurre l'autonomia delle Regioni, diminuendo le loro capacità e potenzialità economiche. Ciò è più difficile da accettare, signora Presidente, se si osserva che il taglio economico non riguarda solo importi e cifre, ma indica - se il testo non verrà modificato come auspichiamo - anche dove tagliare, su quali capitoli, su quali attività, senza tenere conto delle specificità, del tipo di vita della gente che vive in montagna, senza tenere conto di come queste Regioni in passato abbiano speso le loro risorse, se cioè le hanno sprecate o le hanno usate in modo corretto;

I rami secchi, che tutti siamo d'accordo a tagliare e recidere, non sono gli stessi in tutto il Paese. Vorremmo essere noi a decidere di quali servizi privarci.

7. Ciò vuol dire che questo ente storico ed efficiente non avrà i soldi per pagare i guardaparco; ciò vuol dire impedire a quell'ente di svolgere la sua attività, e questo assume rilevanza non solo per i valdostani, ma per tutto il Paese. Inoltre, i tagli previsti da questa manovra arrivano in un periodo in cui la Valle d'Aosta sta trattando con il Governo il decreto attuativo della legge n. 42, e quindi dei nuovi rapporti economici

mentre si discute a questo tavolo comune, si interviene prescindendo da quel tavolo e da quelle discussioni, abbassando dall'esterno una scure su questa trattativa. Le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta a larga maggioranza - compresi anche alcuni rappresentanti di forze dell'attuale maggioranza di Governo - hanno siglato una mozione che richiede al Governo un intervento di rispetto istituzionale verso la nostra autonomia speciale, e questo in un momento in cui tutti vedono nel federalismo fiscale la soluzione amministrativa più corretta per tutti i problemi del nostro Paese. Ma se l'attuazione del federalismo fiscale, che tutti auspichiamo, si presenta come un percorso forse ancora lungo da attuare, non si può non avvertire come questa manovra costituisca una fermata improvvisa. se questo decreto può essere accettabile nel desiderio di sanare i conti pubblici, con questa metodologia però tutto diventa possibile: tutta la storia, gli accordi in atto, le norme costituzionali, gli Statuti speciali, tutto si potrà modificare in modo unilaterale,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, come è spesso accaduto dall'inizio della legislatura, ci troviamo a svolgere un dibattito un po' surreale. Stiamo discutendo della manovra sin dal 22 giugno scorso, eppure non sappiamo ancora quale sarà il testo che dovremo votare in Aula. E questo accade semplicemente perché profonde sono state e sono tuttora le divisioni interne al centrodestra. Cosa questa che costringerà il Parlamento al 34 voto di fiducia. La cartina di tornasole delle vostre divisioni e del conseguente ricorso al voto di fiducia è rappresentata dal fatto che non accetterete sicuramente la proposta avanzata questa mattina dal senatore Giaretta, nella sua bella relazione di minoranza, di rinunciare al voto di fiducia in cambio di una riduzione a soli 25 degli emendamenti del Partito Democratico. Entrando nel merito del provvedimento, come ormai è stranoto a tutti, quello che contestiamo non è certo la manovra in quanto tale, ma la sua inadeguatezza. Questo Governo continua a non rendersi conto della gravità della situazione in cui versa il Paese. Proprio pochi giorni fa l'ISTAT ci ha ricordato che il tasso di disoccupazione in Italia è arrivato all'8,7 per cento, mentre nel Mezzogiorno supera il 14. Il numero degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni ha raggiunto il 37,7

I giovani rappresentano il futuro del Paese ed un Governo responsabile avrebbe utilizzato la manovra come un'occasione per garantire ai nostri ragazzi quelle opportunità che oggi non riescono a trovare. nel testo che ci viene proposto mancano completamente politiche di sostegno alla crescita che accompagnino il Paese fuori dalla crisi; politiche in grado di promuovere un'occupazione stabile ed il sostegno dei redditi, specie quelli più bassi; politiche che rimettano in moto la domanda interna, che aiutino le imprese in difficoltà nel ricorso al credito e che pianifichino scelte strategiche di politica industriale, di cui l'Italia ha un grande bisogno. Poi ci vogliono le riforme: penso, in particolare, a quella degli ammortizzatori sociali, che il Ministro del lavoro si ostina ad impedire, ignorando che è proprio nei momenti di crisi che sono necessarie riforme profonde per attrezzare il Paese alla ripresa. Peraltro, fra qualche settimana comincerà a scadere per migliaia di lavoratori la cassa integrazione, e nessuno sa cosa accadrà, visto che in questa manovra non c'è un euro. Questa manovra invece propone soltanto una serie di tagli indiscriminati, perché il suo unico scopo è quello di fare cassa, senza dare una prospettiva di ripresa al Paese. Ci si accanisce contro i più deboli proprio quando i più deboli andrebbero maggiormente aiutati e, ovviamente, si salvano "lor signori", a conferma di uno degli *imprinting* di questo Governo. Basti pensare che addirittura il 90 per cento dei tagli previsti da questa manovra pesa su Comuni, Province e Regioni, mettendo così a rischio servizi essenziali per i cittadini. Lo stesso vale per i tagli alla previdenza, che rappresentano un vero e proprio ladrocinio ai danni di chi ha lavorato una vita intera; ladrocinio che si compie con il pieno consenso del Ministro del lavoro. Questo è esattamente, purtroppo, un altro segno dei tempi. E non mi riferisco alla beffa del famoso refuso; penso invece al fatto che comunque la norma sui 40 anni di contributi è stata cancellata, perché, come per i 60 anni per le donne e i 65 anni per gli uomini, dall'anno prossimo bisognerà lavorare un anno in più. Faccio notare che, nel caso dei 40 anni di contributi, ciò significa che la lavoratrice o il lavoratore pagheranno un anno di contribuzione senza che la propria pensione aumenti di un solo euro. Il ladrocinio si completa con il fatto che il prodotto di questi tagli non resterà nel sistema previdenziale, ma verrà letteralmente scippato per essere incamerato dalle casse del ministro Tremonti. Non era mai successo prima. A questo proposito, vorrei sollevare anche una questione con cui questa maggioranza non ha particolare dimestichezza: parlo, in generale, del rispetto delle regole e, nello specifico, di quelle che riguardano il corretto rapporto fra Esecutivo e forze sociali. Mi riferisco all'accordo del 2 luglio 2007, sottoscritto dal Governo Prodi, da tutti i sindacati, da tutte le associazioni imprenditoriali e confermato da oltre 5 milioni di lavoratori con un *referendum*. Un accordo cancellato da voi con un atto unilaterale, senza consultare le parti sociali. Allo stesso modo, la manovra recepisce acriticamente la normativa europea che impone di portare a 65 anni l'età pensionabile delle donne. Il Partito Democratico propone saggiamente di ritornare allo spirito della riforma Dini, introducendo qui una maggiore flessibilità nel sistema pensionistico. Ma voi non sapete di cosa si parla. C'è poi il capitolo dei tagli al pubblico impiego. Parliamo di semplici lavoratrici e lavoratori che guadagnano in media 1.200 euro al mese. La manovra di fatto blocca la contrattazione, anche qui violando regole precise sulla sovranità delle parti nel negoziato, punendo una categoria non certo privilegiata, mentre non si chiede alcun sacrificio a chi ha disponibilità economiche infinitamente maggiori. Ma, come dicevo, questi appunto sono "lor signori". Si reitera il blocco del *turnover,* la riduzione delle risorse per i contratti a tempo determinato, per i co.co.co., per i co.co.pro. e per gli interinali, con il risultato che moltissimi precari saranno mandati a spasso. Si infligge l'ennesimo colpo alla ricerca scientifica, che invece costituisce la pietra angolare delle politiche economiche di tutti i grandi Paesi. Per risparmiare qualche euro, il Governo cancella con un colpo di spugna enti di eccellenza, come l'ISAE, il cui torto non è certo quello di lavorare con grande professionalità, competenza ed autonomia, bensì quello di aver fatto qualche previsione di politica economica non esattamente collimante con quelle del Ministro dell'economia. Si cancella, per le ragioni che ha esposto giustamente il collega Casson, l'ISPESL. Presidente, consegnerò poi il testo del mio intervento. La crisi sta cambiando profondamente il mondo in cui siamo abituati a vivere. Le certezze della mia generazione e di quella precedente, le idee novecentesche di una crescita continua, di un benessere destinato naturalmente ad aumentare con il passare degli anni, di un lavoro stabile in un'azienda fino alla pensione sono state cancellate. I ragazzi di oggi hanno paura del futuro; la precarietà rappresenta ormai drammaticamente una condizione di vita. Questa crisi ha avuto il merito - se così si può dire - di far capire a tutti che è arrivato il momento di cambiare e che questo modello di sviluppo non è più sostenibile. L'euforia verso il liberismo e la finanza, verso la mano invisibile del mercato come soluzione a tutti i problemi si è sciolta in un attimo nell'estate di due anni fa. La politica oggi ha il compito principale di non ripetere gli errori del passato; ma per fare questo bisogna investire, come saggiamente fanno i nostri *competitors* internazionali, non tagliare e basta, perché dalle scelte che facciamo oggi dipenderà il nostro futuro. Onorevoli colleghi della maggioranza, sinceramente non riesco a capire quale futuro il Governo abbia in mente; forse perché, semplicemente, un'idea di futuro questa maggioranza non ce l'ha. *(Applausi

il risanamento del debito pubblico, che è un problema dell'economia e della politica italiana da almeno un quarto di secolo, e che oggi rappresenta un vincolo aggiuntivo particolarmente stringente, poiché abbiamo un debito pubblico *pro capite* di oltre 30.000 euro - quindi tra i più alti del mondo - a fronte di un debito privato inferiore a quello di tutti i Paesi sviluppati. è un vincolo per una manovra che invece ha un altro obiettivo: dare una risposta alla più grave recessione degli ultimi decenni ed aiutare una ripresa per niente scontata. Non è vero, tra l'altro, che la globalizzazione trascina tutti insieme verso la ripresa, perché i Paesi meno competitivi questo non lo vedranno, o lo vedranno con enorme ritardo rispetto agli altri. L'obiettivo di questa manovra non è dunque il risanamento, quindi la ripresa, quindi la crescita, quindi la competitività. Il *World Competitiveness Scoreboard* del 2010 ci dà in risalita, ma al quarantesimo posto nel mondo e al ventesimo posto in Europa per competitività. Di per sé, ridurre la spesa pubblica non è uno strumento di crescita. (il periodo di Keynes e e Roosevelt), proprio l'aumento della spesa pubblica è stato ritenuto lo strumento per eccellenza per sostenere la domanda aggregata e far ripartire l'economia. Allora si trattava soprattutto di investimenti in grandi opere pubbliche, nelle infrastrutture, nel *welfare*. Oggi molte cose sono cambiate e si è capito che l'aumento incontrollato della spesa pubblica genera inefficienza, monopoli, occupazione partitica dell'economia. pertanto aggredire le sacche di spesa improduttiva, le rendite monopolistiche, le incrostazioni corporative che si annidano sia nell'apparato pubblico sia nelle interazioni spesso collusive e talora addirittura criminali che esso ha con componenti deviate del comparto privato. Ciò che bisogna colpire non è però la spesa pubblica in quanto tale, ma la sua improduttività. sostituire gli sprechi, che sono quasi sempre pubblici perché pagati con soldi altrui, con investimenti, pubblici o privati, che siano capaci di generare economie esterne, competitività, ad esempio nei trasporti, nella ricerca, nella formazione, ciò richiede misure strutturali, come ad esempio - e non ce n'è traccia, purtroppo - lo smantellamento del costosissimo e clientelare capitalismo municipale, ossia il castello di scatole cinesi con cui i Comuni gestiscono servizi che potrebbero tranquillamente acquistare sul mercato. Detto ciò, il giudizio è difficile, come ho già precisato. Questa manovra è per molti aspetti coraggiosa, perché aggredisce quei gangli in cui si annida lo spreco pubblico, e in qualche caso lo fa finalmente senza riguardo per gli interessi corporativi che si sono stratificati negli anni della malapolitica. Essa affronta il rischio di impopolarità come raramente si era usato in passato. per la ripresa ci sarebbe stato probabilmente bisogno di più riforme per ridare competitività ed attrarre investimenti anche internazionali. Alcune sono in corso: dalla riforma dell'università, al rilancio del nucleare, al federalismo, alla rivoluzione dei rapporti tra l'impresa, la libertà di impresa e la sua utilità sociale. Altre purtroppo, anche se presenti nel programma del Governo, sono oggi un po' al al palo, come le liberalizzazioni cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. Nel frattempo, nel breve periodo, non si può prescindere dai tagli agli sprechi, sapendo però che il taglio alla spesa e ai consumi di per sé non fa ripartire l'economia, anzi la può

I tagli orizzontali non sono quasi mai intelligenti e tanto meno meritocratici. Il Comune formica, che ha già tagliato negli anni passati, non può essere colpito come il Comune cicala che non lo ha fatto. È più facile, però è sbagliato ed è anche diseducativo, come un po' accade Si poteva cogliere l'occasione forse per traguardare un costo standard dell'amministrazione comunale. Si poteva fare altro; si poteva entrare nel merito della montagna di acquisti delle pubbliche amministrazioni, senza aver troppa paura di danneggiare quella parte dell'economia privata che si arricchisce con risorse pubbliche approfittando di meccanismi di spesa che non sono né trasparenti né concorrenziali. Si potevano introdurre sistematiche valutazioni del merito dei dipendenti pubblici di tutti i comparti, inclusi quelli che operano dietro il paravento di società di diritto privato, con i loro *grand commis* dai redditi milionari. Si potevano monitorare gli sprechi delle fondazioni bancarie, che si stanno sempre più sostituendo alle amministrazioni locali nel gestire quantità ingenti di risorse dei territori in cui si trovano. i settori che secondo la disattesa Agenda di Lisbona dovrebbero essere quelli su cui un'economia moderna e competitiva costruisce il proprio futuro. E non lo stiamo facendo, come altri Paesi europei per la verità. Con questi tagli, altro che rientro dei cervelli! Nel momento in cui abbassiamo o congeliamo la retribuzione dei giovani professori e dei ricercatori con danni di decine, forse centinaia di migliaia di euro ma per contro manteniamo uguale lo stipendio di tutti loro, quelli bravi e quelli cattivi, diamo loro un messaggio preciso: a quelli bravi diciamo che se ne possono restare all'estero perché hanno tutto l'interesse a farlo; a quelli cattivi diciamo che possono restare qui perché la loro mediocrità non sarà certo un ostacolo, anche perché nel frattempo i migliori saranno andati via. E poi si doveva mettere mano alle misure fiscali

non tanto rinunciando invece alle garanzie liberali del contenzioso tributario per il cittadino o per la piccola impresa, che viene colpita magari da una sanzione errata dell'amministrazione tributaria, mentre poi leggiamo che il 47 per cento degli inquilini estivi di Porto Cervo continua ad essere formato da nullatenenti. non è sbagliata l'entità quantitativa della manovra, nemmeno la sua strategia, ma si poteva e forse si doveva fare meglio per renderla più intelligente e quindi utile alla competitività del Paese, per favorire la ripresa, perché questo è l'obiettivo del provvedimento, e non solo il risanamento dei conti pubblici ottenuto in qualunque modo. Anche per questo considero negativo aver posto per l'ennesima volta la questione di fiducia. So che in altri Paesi le manovre di bilancio sono blindate anche per Costituzione. Qui però abbiamo perso un'occasione per migliorare questa manovra. Per usare un paradosso usato qualche volta dal presidente Obama, non dovevamo sprecare una crisi così seria da permetterci di fare cose che prima non avremmo mai potuto fare. Detto questo, stiamo comunque dando al Paese ed all'Europa un importante segnale di serietà e di rigore. È in fondo il primo grande segnale dopo molti anni di inerzia, e questo è forse il motivo principale, oltre - lo ammetto - alla disciplina di partito,

voglio denunciare, anche se in un'Aula praticamente vuota, il grande assente dalle pagine che descrivono questa manovra: un grande assente chiamato futuro. Ed è assente non solo perché manca completamente la previsione di un qualsiasi strumento atto a favorire la ripresa economica e sociale del nostro Paese, ma manca il futuro, perché mancano interventi per far fronte alla drammatica situazione in cui versano le giovani generazioni.

più del triplo del tasso di disoccupazione nazionale. Il 63 per cento degli occupati, invece, è vittima della cosiddetta flessibilità del lavoro, e proprio sui giovani cosiddetti flessibili

Questo dato conferma dunque che, in Italia, un giovane su tre è disoccupato. L'impatto della crisi sull'occupazione ha quindi trovato un ammortizzatore sociale gratuito. Ha colpito un bersaglio molto facile: ha colpito prede intrappolate in rigide gabbie che impediscono quella mobilità sociale di cui hanno usufruito le generazioni precedenti, precedenti, immobilizzate nell'impossibilità di progettare il proprio domani, indebolite dalla precarietà, da salari - ove presenti - bloccati da quindici anni e dall'assenza totale di tutele e di garanzie. L'iniquità intergenerazionale è la più grande ingiustizia sociale dei nostri tempi. Questo processo avanza in modo inesorabile. Due milioni sono i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Di questi, circa la metà non cerca impiego, nella convinzione che quella ricerca non servirebbe a nulla. Il blocco della visione di prospettiva è ormai stato interiorizzato nella gran parte dei giovani. Siamo quindi di fronte alla formazione della più imponente, nuova e inedita categoria, completamente al di fuori dalle categorie tradizionali a cui ci eravamo abituati nel Novecento e nei primi anni di questo millennio, che in modo silenzioso, ma molto veloce continua ad implementare le proprie fila. Sono un esercito di invisibili, immobili e inattivi giovani uomini e giovani donne a cui è negato il futuro, privando, di conseguenza, di futuro il nostro Paese. Sono invisibili per chi dovrebbe preoccuparsi ed occuparsene, ossia chi oggi decide le politiche nazionali ed è nelle condizioni di affrontare quei dati che ormai sembrano dei bollettini di guerra. Chi governa non solo non li rende attivi e non se ne preoccupa, ma pare proprio che non se ne voglia occupare anche per i prossimi due anni. Le conseguenze sono la grave e persistente iniquità, il blocco della crescita del nostro Paese e una società che continua a invecchiare in modo inesorabile. Questo è il più grande dramma individuale e collettivo del nostro Paese e del nostro tempo e l'effetto depressivo e recessivo della manovra, negandolo, lo procrastina in modo inesorabile per i prossimi anni. L'effetto delle ristrettezze delle risorse e delle tutele, senza misure di supporto alla crescita, caricherà sulle spalle delle giovani generazioni il peso più grande della crisi economica. L'indifferenza con cui il Governo, nonché la maggioranza che lo sostiene, affronta questo dramma è assoluta. Non un euro delle maggiori entrate previste sarà impiegato per affrontare questa emergenza. Anzi, molti dei tagli alla spesa prevista aggraveranno ulteriormente le condizioni delle nuove generazioni: i pesanti tagli alla scuola, il probabile taglio dei contratti temporanei nella pubblica amministrazione, i tagli agli enti locali titolari delle politiche attive del lavoro, delle politiche sociali, delle politiche di sviluppo territoriale non faranno altro che gravare sui giovani, sulla ricchezza e la fantasia che solo le nuove leve le nuove leve sono in grado di proporre e sulle possibilità di crescita del nostro Paese. Tutto ciò si è inserito poi nelle scelte che questo Governo ha già fatto nei due anni precedenti, che abbiamo trascorso senza alcuna attenzione per le nuove generazioni, e che hanno sicuramente inciso su un quadro così preoccupante, che colloca l'Italia in una situazione di primariato nella crescita dell'esercito dei «senza futuro». Gli altri Paesi, che pur non hanno i valori della disoccupazione giovanile pari a quelli dell'Italia, hanno fatto scelte diverse: nessuno ha tagliato fondi alla scuola, all'università, alla ricerca. Anzi, di fronte a manovre anche di dimensioni superiori hanno impostato scelte di investimento composte da elementi fortemente innovativi.

per i giovani, che avevamo chiamato Piano straordinario per l'accesso all'autonomia finanziaria delle nuove generazioni: un intervento di 5 miliardi che avevamo indicato venisse finanziato con una riduzione delle risorse assegnate ai singoli Ministeri, che sono i meno interessati agli obiettivi di risparmio di questa manovra. Già non abbiamo ottenuto alcuna considerazione in Commissione, e l'indicazione della fiducia a chiusura di questo provvedimento ci dice che probabilmente nulla cambierà nei prossimi due giorni, però il Partito Democratico continuerà a portare avanti la sua battaglia e a denunciare l'assenza di interesse e impegno, cercando con tutti gli strumenti a disposizione di aprire degli spazi di iniziativa che favoriscano politiche a a sostegno dell'autonomia dei nostri ragazzi, ai quali si continua a rapinare il futuro.

suo complesso è ampiamente negativo. Riteniamo che questa manovra finanziaria sia iniqua, squilibrata e soprattutto al di sotto delle esigenze e delle necessità del Paese, anche perché l'assenza di riforme di carattere strutturale ne riduce l'efficacia e ci esporrà sicuramente a degli interventi correttivi in un prossimo futuro.

si è conclusa positivamente, grazie anche al forte intervento in Commissione bilancio che l'Italia dei Valori ha attuato attraverso il suo Capogruppo e grazie anche ad un'iniziativa

che prevedeva che i benefici per le imprese alluvionate si applicassero esclusivamente ai versamenti tributari. Ne parlo perché si tratta di questione che riguarda la mia Regione e che, se non avesse visto un intervento così forte in Commissione, probabilmente sarebbe rimasta così come scritta e proposta dal Governo.

e che, grazie alla legge n. 350 del 2003, si erano viste riconosciute il diritto al pagamento in misura ridotta, in particolare nella misura del 10 delle somme che erano dovute negli anni, dal 1994 in avanti, quindi nel periodo post-alluvione, a titolo di tributi. Poi tali agevolazioni erano state anche estese ai contributi INPS, INAIL eccetera.

È evidente che la proposta che era stata fatta dal Governo nella manovra, volta ad escludere sostanzialmente tali benefici, avrebbe portato queste aziende sull'orlo del collasso.

Invece, purtroppo, nonostante anche in questo caso l'Italia dei Valori abbia presentato un emendamento e un ordine del giorno,

Questo è un altro tema di cui hanno già parlato alcuni colleghi in interventi precedenti che però voglio riprendere. Come tutti sappiamo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro del lavoro ha funzioni importantissime. Voglio ricordare in particolare, essendo responsabile, all'interno della Commissione d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, della Sottocommissione prevenzione e formazione,

funzione istituzionale - dicevo - a cui l'ISPESL da sempre si è dedicato con moltissima attenzione, tanto è vero che ormai da qualche anno portava avanti progetti importantissimi, soprattutto nel settore scolastico (in particolare nella scuola primaria e secondaria), ed era diventato *task leader*

che avevano proprio l'obiettivo di creare una cultura della formazione e della prevenzione sin dalla scuola primaria. È evidente che la soppressione dell'ISPESL prevista dall'articolo 7 per noi è inaccettabile perché queste funzioni non riteniamo possano essere svolte in modo altrettanto proficuo funzioni, così come previsto dal disegno di legge. Crediamo, quindi, che questa scelta sia oggettivamente incomprensibile e vada comunque a detrimento della lotta agli infortuni sul lavoro che credo

che sia garantita l'indipendenza dell'ISPESL e la continuità del pieno esercizio di tutte le sue funzioni, che siano salvaguardate tutte le professionalità attualmente in servizio e, soprattutto, che siano salvaguardati tutti i progetti di ricerca che l'ISPESL molto bene sta portando avanti.

(come è stato peraltro ricordato anche in uno degli ultimi interventi da un esponente della maggioranza che ha detto molto sinceramente che voterà questa fiducia

che non consente, ancora una volta, a quest'Aula, e non consentirà, verosimilmente, neanche alla Camera di apportare dei miglioramenti a delle misure economiche comunque gravose che, come al solito (da oltre due anni a questa parte, da quando si è insediato il Governo Berlusconi), guardano sostanzialmente ai tagli e non a uno sviluppo competitivo per il nostro Paese. *(PD)*. Signora Presidente, la forma è sostanza e, evidentemente, anche la forma di questo dibattito non può non essere argomento Dibattito che, come si è ripetuto in quest'Aula in queste ore, dovrebbe decisamente appassionarci tutti. le aule deputate, i luoghi istituzionali, l'Aula del Senato e la Commissione bilancio del Senato, in realtà, non sono i luoghi in cui si dibatte e si decide questa manovra finanziaria, che si decide altrove. Si decide altrove il contenuto, si decidono altrove i criteri e le priorità. Questo è un peccato, perché, probabilmente, io e il senatore Musso avremmo potuto dibattere e trovare anche punti di accordo in quest'Aula. Siamo seduti su lati opposti, eppure, se si fosse dibattuto, forse avremmo trovato molti punti in comune su cui poi andare a incidere per fare una manovra

È una manovra, però, quella che almeno finora abbiamo visto che, in realtà, fa dei tagli lineari il principio su cui si fonda e

dalla lotta all'evasione fiscale, e già questo è un punto grave della manovra.

Del resto, dal lavoro al *welfare*, dalle pensioni alle liberalizzazioni, anche il primo decennio degli anni Duemila è trascorso - con la sola, incompiuta eccezione della legge Biagi - senza quelle riforme strutturali di cui il Paese ha bisogno per interrompere quel che a non pochi appare ed è temuto come uno strutturale, istituzionale degrado o almeno declino. Un declino che per ogni individuo si traduce in minore libertà e responsabilità e, per i più, in maggiore povertà, in minore benessere. Le ideologie hanno continuato ad essere gli alibi all'ombra dei quali hanno ripreso «naturalmente» a regnare corporativismi, assistenzialismi, rendite di posizione, capitalismi di Stato e privati - inquinati dai conflitti d'interesse e drogati dalla spesa pubblica clientelare. Ci si è lasciati governare da fatti e misfatti, invece che governarli. Si sono creati dei tabù e li si è usati come alibi per negare la stessa esistenza di problemi evidentissimi da quasi un mezzo secolo.

La manovra finanziaria presentata dal Governo prosegue, purtroppo, lungo questa traccia: nessuna misura strutturale, tagli lineari, interventi emergenziali, settoriali o a colpi di *una tantum*. Misure inique, dunque, dall'efficacia limitata, ma soprattutto senza alcuna prospettiva, per il nostro Paese, di riforme, crescita, sviluppo. Per distribuire ricchezza, bisogna prima produrla; in caso contrario si distribuisce solo povertà, se non, addirittura, miseria oppure favori e quindi clientelismo. Le iniziative politico-parlamentari che abbiamo promosso come radicali, e che abbiamo tradotto in emendamenti e ordini del giorno - in realtà tutto il tempo preso dalla Commissione bilancio non è certo servito a discutere nel merito emendamenti e ordini del giorno - cercano di ribaltare l'impostazione della partitocrazia, andando a incidere in modo strutturale proprio in quei settori che i conflitti di interessi, i veti incrociati, le difese di rendite di posizione corporative hanno ormai condotto alla disastrosa condizione

A quel punto si sarebbe dovuto ben parlare di *voucher* universali e quindi rivedere e rivoluzionare il concetto dei servizi di cura e di assistenza. delle liberalizzazioni: dal monopolio dell'INAIL alla rete del gas, ai libri, agli sconti, alla vendita dei quotidiani e dei periodici, alle vendite sottocosto (siamo ancora un Paese in cui esistono norme che vietano le vendite sottocosto, gli sconti)

evidentemente fino ad oggi non si è voluto toccare: il finanziamento pubblico ai partiti. Con un nostro emendamento si anticipava al 1° gennaio 2011 la riduzione del 10 per cento del finanziamento pubblico ai partiti,

municipalizzate alla razionalizzazione dei trasferimenti finanziari, alla fiscalità ambientale. Tanti potevano essere gli argomenti di dibattito, dibattito, tanti gli spunti che potevano arrivare da quest'Aula, ma evidentemente si decide di governare con altri sistemi e, del resto, oggi la pregiudiziale

non con le leggi, senza controlli, senza luoghi decisionali e responsabilità diverse, senza i filtri che la democrazia richiede, ritenuti evidentemente cavilli, cavilli, appesantimenti burocratici da evitare, così come è da evitare questo Parlamento, come luogo in cui discutere le misure e le riforme di cui questo Paese ha urgente necessità. In attesa dell'arrivo del maxiemendamento su cui verrà posta la fiducia, cortesemente ringrazio per la cortesia di avermi fatto parlare.

La domanda è: chi paga per questi conti sbagliati? E, soprattutto, il prezzo pagato - da pochi - sarà sufficiente a presentare l'Italia con i conti in ordine alla valutazione dei mercati internazionali e con le carte in regola nei confronti dell'Unione europea? La nostra valutazione è che entrambe le risposte siano, purtroppo, negative. Nonostante questa assenza di risultato, la manovra pesa, mettendo le mani nelle tasche di molti, soprattutto di coloro verso i quali questa operazione riesce più agevolmente: ceti medi, lavoratori dipendenti, lavoratori della pubblica amministrazione. C'è fra costoro un elemento di diversificazione fondamentale, che valorizza diversamente il peso della manovra: il genere. La Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di valutare l'impatto di genere delle misure anticrisi, considerando il mercato del lavoro non neutro, ma un ambiente in cui uomini, donne, coppie e famiglie hanno un posizionamento diverso. In particolare, secondo l'Europa devono essere valutati la revisione dei sistemi di sostegno al reddito per la disoccupazione, la revisione del sistema dei congedi parentali, l'investimento in infrastrutture sociali. Ciò, a partire dal presupposto che questi elementi operino diversamente rispetto all'opportunità di occupazione delle donne e che l'occupazione delle donne sia fattore fondamentale per la crescita e la competitività dei Paesi. La manovra al contrario, ha un profilo penalizzante per l'occupazione e la condizione economica delle donne. Gli interventi di riduzione della spesa pubblica operano innanzitutto nel settore del pubblico impiego, congelando le retribuzioni, contenendo ad un quinto la sostituzione del *turnover*, licenziando la metà dei precari della pubblica amministrazione. Le donne sono il 55 per cento dei dipendenti della pubblica amministrazione, con punte che arrivano al 78 per cento già pesantemente colpita dagli interventi Gelmini, e del 62 per cento della sanità, dove sono collocati oltre la metà dei posti di lavoro del pubblico impiego

dagli effetti di una politica di risanamento dei conti pubblici basata su una riduzione di quella infrastrutturazione sociale considerata al contrario fondamentale per incrementare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Anche il relatore, senatore Azzollini, ha definito obiettivo fondamentale per la ripresa della crescita l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro. Noi riteniamo che un possente elemento di promozione della crescita risieda proprio nell'occupazione delle donne, perciò abbiamo caratterizzato la nostra proposta mettendo in primo piano misure fiscali volte a favorirla: l'aumento delle detrazioni per le spese di cura e per servizi, la «dote fiscale» per i figli, il riordino del *mix* di detrazioni e *bonus* economici per la famiglia, la proposta di riduzione dell'aliquota marginale per la tassazione dei redditi delle donne lavoratrici, dipendenti od autonome, la fiscalizzazione di quota parte degli oneri sociali per le imprese che assumono donne costituiscono un pacchetto di misure non solo improntato alla redistribuzione del reddito, al compito cioè di utilizzare il fisco come strumento di equità, ma anche alla promozione dello sviluppo. Anche il tema delle pensioni è stato da noi affrontato in termini di proposta; anche su questo non abbiamo goduto nemmeno del beneficio del confronto. Possiamo convenire sull'opportunità di una riflessione su temi quali la sostenibilità nel tempo delle pensioni, non solo per il bilancio dello Stato ma anche per la vita delle persone, l'adeguatezza e l'equità del sistema pensionistico pensionistico vigente; certo non possiamo condividere il metodo con cui si è scelto di intervenire, né le soluzioni adottate. Gli effetti di genere delle scelte del Governo sono pesantissimi. La norma che posticipa l'accesso al pensionamento di vecchiaia, anche fino a diciotto mesi dal conseguimento dei requisiti, congelando di fatto il diritto al pensionamento, senza riconoscere alle lavoratrici e ai lavoratori alcun beneficio - né salariale, né pensionistico - per il prolungamento dell'attività lavorativa, colpisce particolarmente le donne, che - come è noto - in relazione al tardivo accesso al lavoro, alla discontinuità delle carriere e della contribuzione, in relazione agli impegni di cura, accedono in via largamente prevalente alle pensioni di vecchiaia, non raggiungendo che raramente i requisiti di anzianità lavorativa. Si dirà: «Ma le donne vivono di più». Statisticamente vero, soggettivamente di difficile sostenibilità, considerando che la qualità della vita dipende anche dalla consistenza del trattamento pensionistico, su cui la norma non ha alcun effetto di miglioramento: le donne saranno chiamate a lavorare di più e gratis. Questo prefigura un modello sociale nel quale la riduzione delle spesa pensionistica porta in prospettiva a pensare a un aumento della spesa sociale per la necessità di interventi su fasce di popolazione - prevalentemente formate da donne e bambini - che in maniera sempre più consistente scivolano verso la povertà. Infine, faccio riferimento

Siamo comunque consapevoli della necessità di adeguarsi alle prescrizioni dell'Unione europea, ma non con l'intervento a senso unico che ha scelto il Governo e che ora viene declinato come proattivo alla costruzione di un *welfare* delle pari opportunità che viene rifinanziato sostanzialmente con le risorse che derivano derivano dalla prosecuzione del lavoro delle donne. Il modello è chiaro: la cura dei figli, l'assistenza ai non autosufficienti è questione delle donne: o la svolgono direttamente o la pagano con le risorse derivanti dal prolungamento del loro lavoro. Tutto questo è inaccettabile! abbiamo avanzato proposte, come quella di recuperare lo spirito e la norma della riforma Dini a partire dal pubblico impiego, proponendo un modello di accesso flessibile all'età pensionabile, abbiamo altresì proposto che alle donne venga riconosciuto pienamente il tempo dedicato alla maternità, alla cura dei figli e all'assistenza, attraverso il riconoscimento della contribuzione figurativa per le maternità e per i periodi di assenza dal lavoro dedicati alla cura. Era una proposta sostenibile; si tratta però, purtroppo, di una proposta che nasce nel segno della responsabilità e dell'equità, e niente, niente, è più estraneo alla manovra in discussione di queste caratteristiche, fondamentali per la coesione e la giustizia sociale.